Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, i tempi sono stati ripartiti tra i Gruppi onde consentire la votazione delle mozioni entro le ore 14 di oggi. Come abbiamo comunicato ieri, anche ai Gruppi singolarmente, abbiamo deciso che introdurrà i lavori l'intervento del ministro della difesa Arturo Parisi, che ringrazio per la sua presenza perché ha dovuto posporre un importante impegno istituzionale, il quale però potrà restare con noi solo una parte della mattinata, mentre saranno presenti per tutta la durata dei lavori il vice ministro Intini e il sottosegretario Forcieri.

le mozioni poste all'ordine del giorno di questa Assemblea, che ci accingiamo a discutere unitamente agli altri atti di sindacato ispettivo, muovono dalla vicenda relativa all'ampliamento della base militare di Vicenza, in concessione d'uso all'esercito degli Stati Uniti nel quadro degli accordi bilaterali con l'Italia all'interno della NATO. A tal riguardo, nel corso degli ultimi mesi il Governo è intervenuto in Parlamento numerose volte. a pochi giorni dall'insediamento dell'Esecutivo, il 31 maggio dello scorso anno il vice presidente del Consiglio Rutelli, in sede di *question* *time*, aveva avuto occasione di dare conto della problematica. A questo primo intervento sono seguite poi, nell'ordine, le informazioni rese il 6 luglio dal ministro per i rapporti con il Parlamento Chiti, il 13 luglio dal sottosegretario per la difesa Verzaschi, il 26 luglio da parte dello stesso Presidente del Consiglio dei ministri, il 27 settembre, in risposta a tre interrogazioni distinte, da parte di chi vi parla e, infine, dal ministro per l'attuazione del programma di Governo Santagata lo scorso 24 gennaio e, nuovamente, ieri 31 gennaio. In ognuno di questi interventi, il Governo ha illustrato sempre una ed una sola linea di orientamento, ripetendo quasi alla lettera la stessa esposizione, che è affidata agli atti parlamentari e che non posso che riproporre negli stessi termini. La linea muove dal riconoscimento dell'esistenza, da parte del Governo americano, di aspettative consolidate, fondate sulla disponibilità manifestata dal precedente Governo, di corrispondere favorevolmente alla richiesta avanzata al riguardo dagli Stati Uniti; questo pur in assenza di impegni compiutamente formalizzati. La formalizzazione di questi impegni era infatti condizionata alla disponibilità di un progetto dettagliato di un piano preciso di transizione sulla tempistica, le azioni da compiere e i relativi costi. Questa era appunto la formula presente nella prima risposta resa alla Camera dal vice presidente del Consiglio Rutelli. Tuttavia, ritenendo non irrilevanti le obiezioni avanzate da parti significative della comunità locale e giudicando di rilievo l'impatto che il nuovo insediamento avrebbe avuto sulla città dal punto di vista urbanistico, sociale e ambientale, il Governo, mentre confermava la compatibilità del progetto con le linee di politica estera e di difesa del Paese, ha ritenuto di procedere alla decisione finale solo sulla base di un pronunciamento esplicito della comunità locale. Questo perché il progetto, pur non modificando la qualità militare dell'insediamento esistente, ne modificava certamente la quantità, con conseguenze sociali, territoriali e ambientali, che riteneva concretamente valutabili solo con il coinvolgimento della comunità locale. Pur nella consapevolezza che la responsabilità ultima della decisione rientrasse comunque nella competenza primaria del Governo, in considerazione della sua attinenza alla politica estera e di difesa, nell'attesa della pronuncia della comunità locale, veniva sospesa la decisione conclusiva. Si procedeva quindi a coinvolgere e sollecitare gli organi di rappresentanza locale, perché esprimessero un giudizio di fattibilità sul progetto di ampliamento stesso, naturalmente per gli aspetti di loro competenza. Tale posizione è stata poi rinnovata in tutte le dichiarazioni rilasciate a margine degli incontri che chi vi parla ha tenuto in questi mesi con le diverse parti coinvolte per illustrare la posizione del Governo: incontri con il sindaco di Vicenza Hullweck, con il sindaco di Caldogno Vezzaro, con una delegazione di cittadini di Vicenza e con esponenti di Gruppi parlamentari che avevano chiesto al riguardo delucidazioni. La reiterazione degli argomenti svolti in questi mesi potrebbe quindi esimere il Governo da ulteriori ripetizioni di posizioni già illustrate e affidate agli atti; il rispetto verso il Parlamento e il dovere di massima trasparenza verso i cittadini, ed in particolare verso quelli di Vicenza, ci impongono, tuttavia, di ripercorrere le diverse fas*i* dell'*iter* relativo alla vicenda. La prima richiesta orientativa da parte degli Stati Uniti perviene al Governo italiano nell'ottobre del 2004: in essa si richiede un'autorizzazione di massima ad utilizzare le infrastrutture e le aree dell'aeroporto Dal Molin, in via di rilascio dall'Aeronautica militare italiana. La richiesta non fa riferimento a progetti di insediamento di nuovi reparti, ma solo all'utilizzo delle stesse aree e infrastrutture da parte delle forze già presenti in quel territorio. Il ministro della difesa, onorevole Martino, informato della richiesta dal Capo di Stato maggiore della Difesa, ammiraglio Di Paola, manifesta il proprio orientamento favorevole, ferma restando naturalmente la necessità di svolgere tutti gli approfondimenti relativi. Nel corso del 2005, gli Stati Uniti, dopo aver individuato con maggior precisione le aree potenzialmente disponibili, perfezionano la richiesta, annunciando, per la prima volta il 22 agosto, l'intenzione di incrementare la loro presenza militare, unificando in Vicenza l'intera 173ª Brigata aviotrasportata e trasferendo quindi, nella stessa base, la parte della brigata dislocata in Germania. Vengono in seguito avviati contatti di natura esclusivamente tecnico‑istruttoria tra le autorità militari americane e la Direzione generale del Ministero della difesa, responsabile del demanio militare e degli aspetti tecnici infrastrutturali. Alla fine del 2005 la Direzione generale del Ministero della difesa conferma la fattibilità tecnica generale del progetto, ferma restando la necessità di giudicare la progettazione di dettaglio che avrebbe dovuto ricevere anche il vaglio delle autorità civili regionali in sede di Comitato misto paritetico Difesa-Regione.

Conseguentemente, l'ammiraglio Di Paola, Capo di Stato maggiore della Difesa, comunica tale disponibilità al Comandante militare statunitense in Europa, con lettera datata 12 dicembre 2005. In quella lettera si afferma, ne do la traduzione in italiano: «Sono lieto si comunicarle la fattibilità della cosa e la disponibilità delle autorità politiche della Difesa italiana a soddisfare la richiesta degli Stati Uniti». La lettera conclude poi: «È superfluo dire che, per la cessione d'uso della citata zona, è necessario prendere in considerazione tutti i dettagli del piano di cessione e formalizzarli nel quadro dell'accordo tecnico che regola l'uso delle infrastrutture nell'area di Vicenza». È sulla base di questa lettera, di questo documento che il Governo americano consolida la propria aspettativa sulla possibilità di realizzare il progetto e procede allo studio di fattibilità dello stesso, che è valutato nel costo di 10 milioni di dollari. Su questa stessa base si fonda lo stanziamento di oltre 300 milioni di dollari per finanziare la prima fase dei progetti nel bilancio difesa per l'anno fiscale 2007, secondo le informazioni rese dall'ambasciatore Spogli con lettera del 24 novembre scorso. A valle della dichiarazione di disponibilità di massima del Governo, di cui alla precedente lettera, nel giugno 2006 il Comitato misto paritetico della Regione Veneto esprime, con un solo astenuto, il proprio parere favorevole sul progetto statunitense. Alla riunione partecipa, in qualità di osservatore, anche il Sindaco di Vicenza. A questo punto, il Governo (siamo ormai nel giugno 2006), riconoscendo la fondatezza delle preoccupazioni manifestate all'interno della comunità locale in ordine alle problematiche relative all'impatto urbanistico, sociale e ambientale indotte dalla realizzazione del progetto, ritiene di dover coinvolgere più direttamente la comunità locale, rappresentata dai suoi organi istituzionali, con l'obiettivo di acquisire un giudizio di fattibilità, fino ad allora mai espresso formalmente in nessuna sede. A tal fine chi vi parla, nel settembre dello scorso anno, scrive una lettera al Sindaco di Vicenza sollecitando un parere formale da parte dell'amministrazione comunale della città. La richiesta peraltro viene confermata anche nell'incontro intercorso con lo stesso Sindaco il 16 ottobre scorso. Il 26 ottobre il consiglio comunale di Vicenza approva un ordine del giorno in cui esprime un "parere favorevole all'accoglimento, nel territorio comunale di Vicenza della 173a Brigata aviotrasportata degli Stati Uniti". L'ordine del giorno approvato pone cinque condizioni che riferisco testualmente, per opportuna conoscenza: assenza di voli militari connessi con l'attività operativa del reparto USA; esonero dell'amministrazione comunale vicentina da ogni onere economico connesso alla realizzazione tanto degli insediamenti quanto delle strutture viabilistiche e delle opportune infrastrutture, compresa la realizzazione di opere esterne all'aeroporto Dal Molin e necessarie all'eliminazione di ogni impatto negativo sul piano viabilistico ed ambientale, ritenute irrinunciabili ad avviso degli enti locali territoriali competenti; assenza di impatti negativi sull'attività dell'aeroporto civile Dal Molin, con totale mantenimento delle sue potenzialità di utilizzo turistico-commerciale; salvaguardia (o realizzazione in altro sito, con onere di spesa a carico dell'amministrazione degli Stati Uniti) di ogni realtà sportiva oggi esistente all'interno dell'area del Dal Molin e soggetta a trasferimento; infine, impegno da parte dell'amministrazione degli Stati Uniti ad autorizzare prioritariamente e preferibilmente risorse professionali locali nella realizzazione delle strutture previste per l'insediamento. Sempre al fine di coinvolgere le realtà locali interessate, il 14 novembre chi vi parla riceve il Sindaco di Caldogno, Comune che confina con Vicenza e coinvolto dal progetto di ampliamento della base americana. Riferendosi alla delibera del suo consiglio comunale del 10 agosto scorso, il Sindaco manifesta la sua preoccupazione in ordine all'inquinamento acustico ambientale, alla sicurezza e alla mobilità, alle infrastrutture e ai servizi. Il Sindaco chiede infine che, qualora l'insediamento militare abbia luogo, il Comune sia coinvolto attivamente nella fase di definizione del progetto stesso. In data 15 novembre, in una seduta straordinaria del consiglio comunale di Caldogno, aperta ai cittadini, queste preoccupazioni e richieste sono confermate in una ulteriore delibera. 17 novembre, a seguito di notizie apparse su «Il Giornale di Vicenza» - e successivamente confermate dalla stessa autorità statunitense - in riferimento ad una *presolicitation notice*, predisposta da organi tecnico-militari americani, tesa ad avviare il progetto di realizzazione delle strutture idonee ad accogliere la 173a Brigata USA, il Ministero della difesa, in una nota di agenzia, dichiara che tale procedura era priva del presupposto essenziale, cioè l'assenso da parte del Governo italiano. Questo in coerenza con la scelta di sospendere la decisione conclusiva fino al completamento dell'istruttoria in sede locale, scelta ha guidato la condotta del Governo, anche in considerazione di notizie relative alla possibile attivazione di un'iniziativa referendaria secondo la normativa prevista dall'ordinamento comunale. Il 14 dicembre, e qui intervengono gli elementi da parte americana, l'ambasciatore statunitense Spogli, da me ricevuto, fa tuttavia presente che la ristrettezza dei tempi parlamentari interni all'ordinamento statunitense rende la risposta da parte del Governo italiano non ulteriormente procrastinabile. Entro il 31 gennaio, ieri, la Casa dei Rappresentanti avrebbe dovuto, infatti, deliberare definitivamente lo stanziamento dei fondi per l'ampliamento della base nell'ambito del piano di ridislocazione delle Forze statunitensi in Europa. Allo stesso modo, l'ambasciatore Spogli, il 10 gennaio scorso, rinnova la richiesta al Presidente del Consiglio, confermando l'urgenza e, quindi, l'indilazionabilità di tale decisione. Il Presidente del Consiglio, dando riscontro alle ragioni dell'urgenza, assicura una risposta tempestiva, una volta sentiti i Ministri competenti. Il 16 gennaio, il presidente Prodi riconosce che i rapporti di amicizia e di cooperazione con gli Stati Uniti impongono una risposta e perciò quella decisione conclusiva che era stata fino a quel momento sospesa. Muovendo, pertanto, dal giudizio di coerenza del progetto di ampliamento con la linea di politica estera e di difesa del nostro Paese, giudizio che ha sempre guidato la linea di condotta del Governo, e considerati altresì i deliberati degli organi di rappresentanza locale, il Presidente del Consiglio ha ritenuto di dover confermare la disponibilità a corrispondere alla richiesta avanzata dagli Stati Uniti. Tale decisione - voglio ricordarlo - è stata successivamente trasferita dal Ministro degli affari esteri al segretario di Stato americano Condoleeza Rice, in un colloquio avvenuto in occasione della riunione dei Ministri degli esteri della NATO tenutasi a Bruxelles il 26 gennaio scorso. A partire da questa decisione, si procederà, pertanto, alla formalizzazione della cessione d'uso delle aree necessarie alla realizzazione del progetto, dopo aver naturalmente considerato i dettagli del piano di transizione, nell'ambito degli accordi che regolano la concessione in uso di infrastrutture agli Stati Uniti nel nostro Paese. In questo quadro, il Governo ritiene suo dovere vigilare affinché le opere che verranno realizzate siano rispettose delle esigenze prospettate dalle comunità locali, con particolare riferimento all'impatto sul tessuto sociale, sulla viabilità e sulle reti dei sottoservizi. Sarà ugualmente dovere del Governo assicurare la massima vigilanza circa il rispetto degli accordi bilaterali in materia di utilizzo della base stessa, per quel che riguarda gli impieghi operativi. Della realizzazione delle opere, così come del loro utilizzo, il Governo terrà informato il Parlamento.

Nella discussione generale sono iscritti i presentatori delle interpellanze e delle interrogazioni. Se qualche interrogante, poiché abbiamo iniziato con le comunicazioni del Ministro, fosse rimasto fuori dalle indicazioni, me lo può segnalare ed io gli darò brevemente

loro presenza, onorevoli senatori, siamo oggi a discutere la mozione che il Gruppo di Forza Italia ha posto all'attenzione di questa Aula del Parlamento per chiarire aspetti inquietanti di politica estera che questo Governo ha trattato con superficialità e ambiguità. Dopo sei mesi si è potuto capire l'*iter* procedurale che il Governo di centro-sinistra ha tracciato su questa vicenda. Soltanto il 30 gennaio scorso il ministro Parisi alla Camera dei deputati ha chiarito quali siano stati i passaggi fondamentali che riguardano l'ampliamento della base militare americana della 173a Brigata paracadutisti di stanza a Vicenza. La base militare di Vicenza è in concessione d'uso all'esercito degli Stati Uniti, nel quadro di accordi bilaterali con l'Italia all'interno della NATO. Il Governo Berlusconi aveva mostrato soltanto disponibilità di massima all'ampliamento nel nel momento della programmazione economica dell'evento da parte degli Stati Uniti. Tutto l'*iter* procedurale viene percorso in questi mesi, quando si è mostrata tutta l'ambiguità di questa maggioranza, la politica dei due forni: da una parte scaricare la responsabilità sui predecessori e in capo alle autorità locali, avendo molta cura di non sporcarsi le mani; dall'altra, timidamente mantenere in vita il rapporto di amicizia con gli Stati Uniti. Una settimana fa anche la Commissione difesa del Senato ha potuto verificare lo stato dei lavori, grazie alla giusta intuizione del presidente della Commissione, senatore De Gregorio. Abbiamo potuto ascoltare le ragioni dei cittadini, ragioni giuste, ragioni, plausibili, che riguardano la *governance* della città. Se la vicenda non fosse stata trattata con ambiguità, si sarebbero potuti trovare soluzioni e rimedi sicuramente apprezzabili dai cittadini. Oggi il clima è esasperato, anche sicuramente da agenti esterni che mirano ad accendere riflettori importanti su posizioni ideologiche estreme e che mirano a mettere in difficoltà questa maggioranza per poi trovare margini di trattativa sulla politica interna. Pertanto, se la politica estera del Governo fosse stata limpida e chiara, non dando corpo alle frange estreme di questa coalizione, oggi a Vicenza si sarebbe potuto discutere sicuramente dei problemi ambientali e urbanistici. Purtroppo, però, in questi mesi si sono dovuti ascoltare i messaggi, a volte rassicuranti, a volte sfuggenti, di questo o quel rappresentante del Governo che interveniva sulla vicenda in ordine sparso a seconda del momento, fino a raggiungere l'apoteosi dell'ambiguità quando il presidente del Consiglio Prodi ha esternato dicendo che la materia non era di sua competenza, ma era soltanto un problema di ordine amministrativo locale. È proprio questo giudizio che lascia perplessi sulla credibilità del Governo nello scacchiere internazionale. Possiamo far credere a Paesi alleati che il nostro Paese non ha una guida stabile, credibile, che non si ha un momento decisionale chiaro? Sarebbe opportuna una chiara e trasparente operazione verità, una verità che dovrebbe chiarire quali siano i rapporti che questo Governo vuol mantenere in ambito NATO. Vogliamo essere protagonisti? A volte, a seconda delle convenienze, delle comparse su questo scenario, ci è sembrato di interpretare, da parte di questa maggioranza, un senso di disgusto alla partecipazione alle varie iniziative internazionali. Noi crediamo nella trasparenza dei comportamenti, nella capacità decisionale del Governo, che dovrebbe dare maggiore impulso ai tradizionali rapporti con gli alleati storici, a mantenere saldi e chiari quali siano i valori culturali, storici e sociali del nostro popolo. Mi auguro, signor Presidente, che questo dibattito possa aiutare il nostro Paese a ritrovare la strada, quella strada che ci ha permesso oggi di essere una nazione che ha rispetto dei diritti civili, umani, che ha come fine la crescita delle popolazioni in stato di disagio e che può permettersi di essere veicolo dello sviluppo dell'umanità.

non credo che serviranno dieci minuti per illustrare la mozione presentata dal Gruppo di Alleanza Nazionale, che nell'impegnare il Governo a riferire in Parlamento ha già ottenuto un primo importante risultato, vista la presenza del ministro Parisi

Il problema peraltro è evidente. Nella nostra mozione la questione non era tanto quella di capire le procedure, né tanto meno di seguire gli atti amministrativi. La nostra mozione è nata in un momento particolare,

ruolo all'interno di questo Parlamento e, come ha dimostrato anche l'intervento del collega Salvi, evidentemente l'opposizione al Governo su questa materia si è trasferita ai banchi della maggioranza.

L'atto che si sta compiendo, l'ampliamento della caserma «Ederle», non è un atto amministrativo, non è un problema che riguarda l'assessore all'urbanistica del Comune di Vicenza e non è una responsabilità del sindaco di Vicenza, anche se se in termini procedurali sembrerebbe così. È un atto che ribadisce, o dovrebbe ribadire, una consolidata alleanza bilaterale, e quindi un rapporto transatlantico tradizionale nella storia della politica estera italiana, vale a dire il rapporto fra l'Italia e gli Stati Uniti. Poiché si tratta di una base americana inserita in una rete di alleanze tradizionali del nostro Paese, quindi anche di quelli della NATO, con questo gesto si vuole ribadire e riconfermare una linea di politica estera propria del nostro Paese. Tutto quanto è avvenuto, sta avvenendo a pochi giorni da una manifestazione, quella che si terrà il 17 febbraio, nella quale una gran parte della maggioranza si riconosce e si ritrova. Si tratterà di una manifestazione di protesta non contro la base di Vicenza, ma contro la politica di alleanza bilaterale con gli Stati Uniti, contro una tradizionale alleanza in nome di un antiamericanismo più volte dichiarato, qualche

sarà nello svolgimento di questo dibattito, sarà negli interventi della maggioranza che noi comprenderemo quello che chiediamo esplicitamente nella mozione, cioè di definire su questo argomento la posizione ufficiale di tutte le forze di maggioranza. Un rapporto bilaterale come quello che ha l'Italia con gli Stati Uniti, infatti, non può essere oggetto di dibattito e di discussione su un tema di questo tipo:

Non discuteremo, allora, dell'ampliamento della caserma «Ederle» di Vicenza, ma discuteremo di un tema importante che è quello delle relazioni internazionali del nostro Paese e delle tradizionali alleanze che hanno segnato la sua storia di questo Paese. Vedete, signor Presidente, signor Ministro c'è anche una derivata importante, che ci ha molto preoccupato, e che è strettamente legata all'immagine che questo dibattito sta dando del nostro Paese sul piano internazionale: non è un caso che il ministro Parisi abbia riferito della garanzia che il ministro degli esteri D'Alema ha fornito al Segretario di Stato alla recente riunione dei Ministri degli esteri della NATO,

che danno credibilità al nostro Paese. È chiaro che a queste relazioni e a questi rapporti sono legate, ad esempio, le nostre presenze in Kosovo, in Afghanistan, in Libano, le nostre presenze militari e politiche in molti scenari di guerra o di costruzione di pace nel mondo intero. Se questa è una scelta legata strettamente alla rete di alleanze che abbiamo costruito, è chiaro che mettere in discussione o contestare questo sistema di alleanze significa togliere credibilità alla posizione delle Forze armate del nostro Paese sui diversi scenari di crisi mondiali. quindi, ed è stato offensivo per il nostro Paese sentir dire dal Presidente del Consiglio che si trattava di un atto urbanistico-amministrativo, come se non si comprendesse che cosa sottende l'opposizione di alcuni partiti di maggioranza all'ampliamento della caserma «Ederle», venduta come una base militare (e non lo trattasse dell'ampliamento di strutture militari nel nostro Paese (e non è così), mentre in realtà tale opposizione è un tentativo di bloccare, limitare, modificare, alterare gli equilibri di un rapporto di alleanze che noi vogliamo solido, confermato, definito e ribadito. quindi, che questo dibattito si svolga con ampia partecipazione, attendiamo di conoscere le opinioni e le prese di posizione che peraltro, attraverso molte delle interrogazioni che sono state presentate, appaiono già molto chiare, perché la maggioranza oggi in quest'Aula ha una grande responsabilità, che è quella di definire e di confermare al nostro Paese che il nostro sistema di alleanze non può e non deve essere modificato e che non c'è nessun atteggiamento nei confronti degli Stati Uniti che sia diverso da quello che ha costruito forti e saldi legami che hanno consentito per lunghi decenni, attraverso queste alleanze, la garanzia della libertà e dell'indipendenza del nostro Paese rispetto al sistema comunista del Patto di Varsavia. È in discussione, quindi, molto di più di un atto amministrativo; è in discussione molto di più di una responsabilità dell'assessore all'urbanistica di Vicenza. Mi auguro che questo dibattito definisca chiaramente queste posizioni e che alla fine di esso vi sia la conferma che il nostro è un Paese credibile, leale e fedele alle alleanze che nel tempo e con grande volontà si è costruito.

di politica internazionale, l'altro è un problema del nostro rapporto di alleanze con gli Stati Uniti - alleanze oltre che cinquantennali che vede le difficoltà di questo Governo proprio al suo interno. Questa è la verità ed essa si evince anche dagli interventi che abbiamo appena ascoltato - il senatore Salvi che ha cercato di intervenire - e sappiamo, signor Ministro, le difficoltà che lei ha avuto e che ha.

di una richiesta di attenzione nei riguardi della popolazione e dei problemi locali per l'insediamento e l'allargamento della base del «Dal Molin».

il vostro Governo, ha il diritto e il dovere di mettere in discussione, se lo ritiene opportuno, ma senza rifugiarsi dietro un parere,

la soluzione che riteniamo ottimale per risolvere il problema dell'insediamento della 173a Brigata al «Dal Molin», cioè l'uso delle strutture

costruire adesso, con un impatto ambientale molto più leggero, con un problema viabile molto più risolvibile.

locali. Ci può essere infatti una soluzione migliore di quella prospettata nel rispetto, ripeto, delle nostre alleanze, che noi sosterremo e sosteniamo, nel rispetto del nostro alleato, ma nel rispetto anche dei cittadini di Vicenza. Questo non è stato fatto, signor Ministro e, con quel rimpallo di lettere fra lei e il sindaco Hullweck, che lei ben ricorda (ho esaminato tutte quante con quella richiesta del pronunciamento, che lei è stato costretto a fare perché spinto dalla sua maggioranza, in quanto non poteva prendere una decisione, ci ha fatto

in quasi 20 milioni di euro l'impatto economico della presenza degli americani a Vicenza.

so che la scelta di concedere in uso un territorio a scopo militare agli Stati Uniti è eminentemente politica, che chiama in causa le alleanze e i trattati internazionali, la collocazione sullo scenario mondiale, le politiche della difesa, i modi per preparare o per prevenire la guerra. Ma ancor più e ancor prima che al Governo che il partito di cui faccio parte sostiene, so di essere qui eletta dai cittadini e dalle cittadine del Veneto che hanno dato il loro voto alla coalizione dell'Unione e Rifondazione Comunista perché trovavano nel programma di Governo riferimenti a un nuovo modo di fare politica, forse anche perché ci hanno trovato l'impegno specifico a tenere la seconda conferenza nazionale sulle servitù militari o perché vi hanno letto il principio sovraordinatore della democrazia partecipata. Invece, queste cittadine e questi cittadini, prima ignorati e umiliati dalle trattative segrete tra il Governo degli Stati uniti e il Governo Berlusconi, dalla complicità del sindaco che oggi ha negato loro anche la possibilità di esprimersi attraverso un *referendum*, *referendum*, ora si sentono traditi dalla decisione del Governo Prodi annunciata alla chetichella a Bucarest, senza nessun ascolto delle loro ragioni, dopo mesi in cui alle nostre richieste di parlamentari dell'Unione si è risposto con bugie o con mezze verità, rassicurando sui tempi lunghi e sull'assenza di vincoli internazionali o militari, delegittimando così i parlamentari e i partiti dell'Unione che in Veneto e non solo si sono sempre pronunciati per il no. Ne fa prova anche l'interpellanza formalmente e tardivamente ritirata solo ieri sera con un *fax* e firmata dalle senatrici Amati, Rubinato e Serafini e dai senatori Treu, Pegorer, Morando, Lusi, Bordon e Nieddu, che si erano pronunciati contro questo progetto considerato anacronistico, pericoloso e insostenibile. È a questi cittadini che, utilizzando il breve tempo concessomi per questo intervento, intendo dar voce in quest'Aula, per far sentire al Governo e a chi ci sente qui e fuori di qui, la loro voce, fino ad oggi inascoltata. Questi cittadini non sono certo antiamericani (Vicenza è nota per essere una delle città più che moderate del nostro Paese), ma avversano questa scelta che considerano antitaliana, perché non rispetta l'autonomia e la sovranità del nostro Paese. Questi cittadini e cittadine chiamano tutte le persone che credono nella pace e nella democrazia a una mobilitazione unitaria il giorno 17. Ci dicono: «Difendiamo la nostra terra per un domani senza basi di guerra». Ascoltiamoli, leggo il loro appello... VANO *(RC-SE)*. Se il Ministro non ascolta, neanche qui i cittadini di Vicenza saranno ascoltati. Credo sia una questione di democrazia seria.

i minuti concessomi in questo dibattito per farle conoscere l'appello che i cittadini di Vicenza, che il Governo non ha mai voluto ascoltare, rivolgono per la mobilitazione del 17. Questi cittadini ci dicono: «Il popolo dei vicentini è contrario alla decisione (...) di concedere il territorio vicentino per la costruzione di una base militare con un impatto ambientale e sociale devastante. La contrarietà è ampia e coinvolge tutti: cittadini, movimenti, sindacati, partiti, associazioni, membri nelle istituzioni ed Enti locali» (coinvolge anche il parere negativo, come lei ha ricordato, signor Ministro, delle amministrazioni comunali di Caldogno e di Dueville). «Sulla base di Vicenza si pongono due questioni: la pace, l'Italia sta facendo passi importanti per restituire all'Europa protagonismo ed autonomia, mentre sul "caso" Vicenza il Governo è in contraddizione con gli atti finora compiuti rispetto alla politica estera e inficia l'esercizio della stessa sovranità nazionale; il rapporto con la comunità locale, la quale non può essere irrisa ma va ascoltata. La politica non può alzare un muro tra se stessa e la comunità. I cittadini devono potersi esprimere e contare». Per mesi Governo e Comune si sono rimpallati la responsabilità della decisione, l'Esecutivo nazionale ha ceduto all'*ultimatum* statunitense: «Il Governo non si oppone alla nuova base Usa», ha sentenziato Romano Prodi e dopo appena due ore migliaia di vicentini sfilavano per le strade del centro cittadino. Vicenza non si arrende alle imposizioni, ha riscoperto quella dimensione comunitaria e popolare che in altri contesti - per esempio a Scanzano Jonico o in Val di Susa - hanno permesso di fermare progetti devastanti. Contro la militarizzazione di una città, contro la costruzione di una base a meno di due chilometri dalla basilica palladiana, Vicenza chiama tutti a «una manifestazione pacifica, di popolo, non violenta e colorata che ribadisce che la democrazia non significa imporre le decisioni dall'alto, ma si costruisce

da chi è deciso ad andare fino in fondo per salvaguardare il proprio territorio, da chi resisterà con tutti i mezzi pacifici, con la politica, con gli appelli, con le mobilitazioni, ma anche con la disobbedienza, con il boicottaggio, con il proprio corpo, a questa scelta che anche noi consideriamo insieme a loro insensata e insostenibile.

Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli senatori, intervengo in questo dibattito nella mia veste di parlamentare vicentino, che ha seguito passo per passo negli ultimi mesi gli sviluppi della vicenda «Dal Molin», e intendo denunciare in questa sede e contestare pubblicamente una gestione maldestra ed irresponsabile da parte del Governo, gestione maldestra ed irresponsabile, che ha finito, in primo luogo, per screditare il nostro Paese agli occhi dell'alleato americano. Mi riferisco, signor Ministro, in particolare alla visita a Vicenza dell'ambasciatore Spogli, che, voglio ricordare, è stato aggredito da un drappello di facinorosi, e difeso soltanto dai vigili urbani del Comune, mentre le forze dell'ordine erano impegnate chissà dove, ed in secondo luogo, e la cosa forse mi preoccupa ancora di più, da parlamentare locale, ha finito per alimentare paure e tensioni, anche sotto il profilo dell'ordine pubblico, nella civile e laboriosa città di Vicenza, che di tutto ha bisogno fuorché di queste tensioni. ha presentato nei mesi scorsi ben cinque atti di sindacato ispettivo sulla vicenda «Dal Molin». Nessuna di queste interrogazioni fino ad oggi ha avuto risposta. Perché fino ad oggi il Governo si è sempre sottratto al confronto parlamentare con l'opposizione e perché a questo dibattito si arriva solo per iniziativa dell'opposizione? In realtà, il Governo ha preferito il muro contro muro, facendo di tutto per alimentare tensioni sia al suo interno, sia a livello locale. Perché lei, signor ministro Parisi, che anche oggi si è vantato di aver ascoltato il parere di tutti, si è invece sempre rifiutato di incontrare i lavoratori civili della caserma «Ederle», che rischiavano di perdere il loro posto di lavoro? I comitati del no sono stati ricevuti in tutta fretta e invece il comitato del sì non è stato degnato neppure di una risposta scritta ad una richiesta di incontro che le era stata formulata. È evidente che, come al solito, per questo Governo e questa maggioranza ci sono figli e figliastri. Sarebbe ora utile per tutti che quelle risposte che non mi sono state fornite nelle scorse settimane potessero essere tratte a conclusione di questo dibattito. Sono convinto, signor Ministro, che da una «operazione verità» sul «Dal Molin», come qualcuno l'ha già ribattezzata, trarrebbe giovamento l'opinione pubblica vicentina, che è ancora frastornata dalla ridda di illazioni e mistificazioni di cui si sono resi protagonisti i mediocri attori del teatrino della politica, ma credo ne trarrebbe giovamento anche l'intera politica nazionale. Non le chiederò, signor Ministro, perché il Governo avesse nei mesi scorsi dichiarato in più occasioni che non esistevano accordi con gli Stati Uniti sanciti dal Governo precedente, che aveva dato solo un assenso di massima, e poi abbia sostenuto che gli accordi invece c'erano ed erano vincolanti, al punto che ad essi non ci si poteva sottrarre. A questo ci stanno pensando già i colleghi della maggioranza, che si sono sentiti traditi, nelle numerose risposte del Governo ai *question time* della Camera, e dal successivo, repentino, ed apparentemente inspiegabile, mutamento di opinione da parte del presidente del Consiglio Prodi. Le chiedo piuttosto, ministro Parisi, perché, dopo aver richiesto con urgenza un parere al Comune di Vicenza, con proprie note formali in data 8 settembre, 15 settembre e 11 ottobre 2006, e dopo che il consiglio comunale di Vicenza si era espresso in data 27 ottobre 2006, lei abbia dichiarato, insieme anche al segretario dei DS Fassino, che bisognava attendere ancora un *referendum* per conoscere l'opinione della cittadinanza. Il Governo ha tentato di scaricare sulla comunità locale una decisione che invece era squisitamente politica e che doveva essere presa a livello centrale, come peraltro lei prima ha riconosciuto. Se, come voi oggi dite, gli accordi raggiunti con gli Stati Uniti erano vincolanti per lo Stato italiano e la colpa di tutto ricade sul Governo precedente, la celebrazione di un *referendum* locale avrebbe forse mutato le cose e avrebbe consentito al Governo di sottrarsi ad un impegno assunto? È evidente che no! Allora, perché non volete riconoscere una volta per tutte che la celebrazione di un *referendum* locale sarebbe stata comunque del tutto inutile e che la decisione del Governo non avrebbe potuto che ispirarsi alla continuità della politica estera e alle esigenze di difesa del nostro Paese? Le chiedo ancora, signor Ministro, perché, dopo il falso *scoop* del settimanale «L'Espresso», che aveva parlato di presenza nella nuova base di sofisticati armamenti ed ordigni e di voli militari dall'adiacente aeroporto, allarmando il sindaco della città e l'intera opinione pubblica locale, nessun esponente del Governo è intervenuto per smentire quell'articolo e rassicurare i cittadini di Vicenza che l'ampliamento della caserma «Ederle» aveva invece carattere semplicemente logistico, trattandosi solo dell'acquartieramento di due battaglioni di soldati e delle loro famiglie? Perché, ancora di recente, il Capogruppo dei Comunisti italiani alla Camera continua a parlare di intenzione statunitense di utilizzare l'aeroporto «Dal Molin» come avamposto da cui far decollare aerei verso obiettivi strategici in Medio Oriente? Come ha commentato un autorevole quotidiano locale nell'edizione di due giorni fa, gettare cherosene sul fuoco della protesta è da irresponsabili. Il presidente Prodi, da Bucarest, il 16 gennaio scorso ha dichiarato che il Governo non si sarebbe opposto all'ampliamento della caserma «Ederle» di Vicenza, in quanto tale decisione non costituiva un problema politico, ma, semmai, solo amministrativo ed urbanistico. È plausibile e serio che una decisione di politica estera e di difesa così delicata venga ridotta dal Presidente del Consiglio al rango di decisione amministrativa? E perché, se di decisione amministrativa si trattava, mai nessun esponente del Governo ha avuto la correttezza e l'onestà intellettuale, dimostrati invece dalla senatrice Lidia Brisca Menapace, che pur milita nel partito di Rifondazione Comunista, la quale, a conclusione di una visita della Commissione difesa del Senato, la scorsa settimana ha pubblicamente dichiarato ai cronisti locali che «il *modus* *operandi* del Comune di Vicenza è stato ineccepibile, nessuno può dire il contrario!»? Io credo, signor Ministro, che queste ambiguità abbiano contribuito a creare quel clima di intimidazione e violenza che si è vissuto nelle ultime settimane a Vicenza e di cui sono rimasti vittima, prima, Franca Porto, segretaria provinciale della CISL, rea di essersi preoccupata della sorte dei dipendenti civili della caserma «Ederle» e, poi, la segretaria provinciale dei DS, Daniela Sbrollini, rea di non aver aderito alla manifestazione del 2 dicembre il consigliere comunale dei DS di Vicenza, Marco Dalla Pozza. Infine, ricordo l'episodio più grave: l'aggressione violenta di cui è rimasto vittima il capogruppo dei DS nel consiglio comunale di Vicenza, Gigi Poletto, a cui voglio manifestare in questa sede la mia personale e democratica solidarietà reo di voler partecipare ad un consiglio comunale che i comitati contrari all'ampliamento della base intendevano boicottare, è stato colpito a pugni nella pubblica piazza da un ex consigliere comunale di Rifondazione Comunista. Ritengo molto grave, signor Ministro, che nessun esponente del Governo si sia preso la briga di condannare questi episodi di violenza e intimidazione e si sia preoccupato di svelenire il clima locale. In realtà, ciò avviene perché, anche su questo tema, l'attuale maggioranza è profondamente divisa al proprio interno e non sa trovare una posizione comune. Allora, la soluzione individuata dal Presidente del Consiglio è stata quella di dire che la decisione era semplicemente amministrativa e che, quindi, di tutto sarebbe responsabile il sindaco di Vicenza. Ma, onorevoli colleghi, vi pare serio tutto questo? Il Presidente del Consiglio finge di ignorare che la materia è sottratta, sia sul piano pianificatorio che procedimentale, alla competenza comunale ed è assegnata in via esclusiva al Ministero della difesa, che è anche proprietario del sito destinato all'ampliamento della caserma,

Vorrei peraltro ricordare al Presidente del Consiglio che il Consiglio comunale di Vicenza ha certamente espresso un parere non negativo all'ampliamento della base statunitense, ma l'ha sottoposto al rispetto di diverse e rigorose condizioni, citate peraltro anche dal Ministro poc'anzi: garanzia di assenza di voli militari dall'aeroporto «Dal Molin»; esonero dell'amministrazione comunale da ogni onere economico connesso alla realizzazione delle strutture viabilistiche ed infrastrutturali; garanzia di assenza di impatti negativi sull'attività dell'aeroporto civile «Dal Molin»; salvaguardia di ogni realtà sportiva esistente *in loco*, in particolare della squadra vicentina di *rugby*; garanzia di impegno dell'amministrazione USA ad utilizzare prioritariamente e preferibilmente risorse professionali locali. Allora chiedo al Governo: cosa ne pensate di queste condizioni? Ritenete di poterle fare proprie nella negoziazione che si andrà ad instaurare con l'amministrazione statunitense? Sarebbe un'occasione sprecata se, a conclusione di questo dibattito, il Governo si dimenticasse di rassicurare la città di Vicenza sul fatto che la decisione di ampliare la base

Riterrei utile e saggio che il Governo organizzasse subito un tavolo di concertazione con gli enti locali e le associazioni dei cittadini, per garantire il minore impatto ambientale dell'insediamento, modificarne, se del caso, alcuni aspetti progettuali e ottimizzare le risorse finalizzate a mitigare i costi sociali. Ho detto che sarebbe utile e saggio che il Governo organizzasse questo tavolo, ma l'esperienza mi insegna - e questo dibattito parlamentare lo conferma - che questo Governo e questa maggioranza non hanno in nessuna occasione dimostrato saggezza e buonsenso. Schiacciati come siete dal peso degli estremisti antiamericani e *no global*, non siete in grado di esprimere alcuna posizione unitaria sulle mozioni di oggi, ma neppure sulla politica estera e di difesa (e questo è ancora più grave per il nostro Paese). Il mio timore è che di questa vostra ambiguità e mancanza di linea politica continuerà a soffrire la comunità di Vicenza, abbandonata a se stessa in questa delicata vicenda, in balia degli estremismi e nell'impossibilità di cogliere le possibili ricadute positive del nuovo insediamento statunitense.

Mi auguro con tutto il cuore di sbagliarmi, nell'interesse della mia città; ma le premesse che oggi sono state poste certamente non mi rassicurano. *(Applausi

*(IU-Verdi-Com)*. Signor Presidente, colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, sono tra quelle senatrici e quei senatori che hanno sottoscritto appelli al Governo perché non concedesse l'insediamento della nuova base militare nell'area Dal Molin a Vicenza e che hanno consegnato al Governo, insieme al mio Gruppo, oltre 15.000 firme di cittadini vicentini contrari al progetto. Invece, il presidente Prodi ha annunciato che non si opporrà alla nuova base USA; questo non solo ha determinato una reazione molto negativa delle popolazioni interessate, ma pone anche a noi, coalizione dell'Unione, un grave problema di merito e di metodo al nostro interno. Per ribadire le ragioni contrarie dei Verdi, dopo aver ascoltato - ovviamente - l'intervento del ministro Parisi, vorrei usare tre argomenti. In primo luogo, il Governo sostiene che questa scelta è coerente con la politica estera e di difesa del nostro Paese. Ma quanto sta scritto nel programma dell'Unione per le nuove politiche di difesa indica una strategia diversa sulla questione basi militari. C'è scritto - leggo testualmente - che «in questo quadro reputiamo necessario arrivare ad una ridefinizione delle servitù militari che gravano sui nostri territori, con particolare riferimento alla basi nucleari. Quando saremo al Governo daremo impulso alla seconda conferenza nazionale sulle servitù militari... al fine di arrivare ad una soluzione condivisa che salvaguardi al contempo gli interessi della difesa nazionale e quelli altrettanto legittimi delle popolazioni locali».

Allo stesso modo, dovremmo avviare un confronto sulla politica estera - c'è scritto nel programma - e sulle politiche di difesa nell'ambito delle alleanze internazionali, senza assecondare ciecamente una nuova base USA, che sembra essere una «postazione avanzata centrale delle nuove guerre contro Africa e Medio Oriente», mentre affermiamo di voler essere saldamente ancorati all'Europa. Questa, e prevalentemente questa, è la ragione principale per i Verdi di opporsi alla nuova base USA, per contrastare la corsa agli armamenti per lavorare attivamente ogni giorno a preparare la pace, contro tutte le guerre. Secondo argomento. Tra le preoccupazioni forti della popolazione c'è naturalmente l'impatto urbanistico ed ambientale sul territorio di Vicenza e dei suoi dintorni:

Ma purtroppo, essendo un'area USA usata per scopi militari, nessuno strumento concreto è stato in grado di assicurare, almeno fino ad oggi, una valutazione ambientale accurata degli impatti diretti ed indiretti del progetto. Ed allora, dato che il ministro Parisi il 26 luglio 2006 inviò a diversi senatori e senatrici (tra cui anche io) una lettera in cui assicurava testualmente che «il Governo intende riconsiderare con gli Stati Uniti il progetto nel suo complesso» ed approfondire le «problematiche relative all'impatto ambientale dell'insediamento, con particolare attenzione all'eventuale saturazione urbanistica ed ai possibili livelli di inquinamento», voglio chiedere: perché questa riconsiderazione e queste valutazioni non sono stati effettuati e perché comunque, in assenza di queste, il Governo Prodi ha dato ugualmente il via libera al progetto? Abbiamo peraltro studiato accuratamente la normativa italiana ed europea in materia di valutazione di impatto ambientale, che esclude le opere di difesa nazionale da questo obbligo. che questa nuova base Usa possa essere ricompresa in tale categoria e quindi riteniamo dovrebbe essere sottoposta a VIA secondo le nostre procedure e secondo le direttive, che stabiliscono per insediamenti con queste caratteristiche una valutazione effettuata su scala regionale. Su questo specifico punto, anche su questo, ci aspettiamo risposte dal Governo e facciamo presente che sarebbe anche un modo molto concreto per consentire a tutti i cittadini di poter partecipare e di avere l'opportunità di avanzare nelle sedi istituzionali le proprie obiezioni al progetto. Vengo al terzo punto, delicatissimo: il problema del coinvolgimento delle istituzioni e delle popolazioni locali. Il ministro Parisi ha spiegato come il Governo - e lo ha ribadito anche in quest'Aula - abbia atteso un pronunciamento delle istituzioni locali con la richiesta di un parere formale: atto doveroso naturalmente, anche se vorrei sottolineare - se mi è permesso - che nel caso del Mose il Governo non abbia rispettato le richieste avanzate con eguale efficacia istituzionale dal Comune di Venezia. Questa però è solo una battuta polemica. In realtà, il problema è che anche il Comune di Vicenza non autorizza l'opera sulla base delle ordinarie procedure urbanistiche (proprio per le sue caratteristiche strutturali); opera su cui come ho già detto non è stata effettuata una valutazione ambientale e su cui il Comune ha deciso proprio ieri di non effettuare un *referendum* proprio perché si ritiene «incompetente». E' evidente il gioco dei rimpalli e delle responsabilità tra Comune e Governo, che ha esasperato e deluso i cittadini e devo dire anche noi. Ma qui il centro-sinistra, e lo chiedo al «mio» Governo, dovrebbe mettere in campo la propria cultura e la propria storia - direi anche la propria differenza rispetto al centro-destra in cui la partecipazione è un valore, in cui i *referendum* consultivi sono uno strumento di ausilio delle decisioni, in cui si cerca una sintesi tra interessi generali ed interessi locali, evitando di metterli in contrapposizione e scommettendo sull'intelligenza dei cittadini di capire e di distinguere. Penso sia proprio per questi valori che l'Unione di Vicenza si è schierata compatta contro il progetto ed adesso è stordita dalla decisione del Governo e dal metodo utilizzato. Sono le stesse ragioni di metodo per cui abbiamo contestato la legge obiettivo per le grandi opere, che come Unione ci siamo impegnati a modificare. Penso, immagino, che con questa decisione il Governo ritenga evidentemente evidentemente di interpretare la volontà della maggioranza del proprio elettorato; ma allora perché non consultare il proprio elettorato come già è stato fatto egregiamente con le primarie dentro l'Unione per la scelta del candidato *Premier* e vedere poi quali risultati

i problemi politici che una decisione come questa comporta, per esempio su quale scala effettuare il *referendum* consultivo tra i cittadini o come pesare l'interesse locale con quello nazionale. Sono problemi istituzionali molto delicati e difficili, ma il Governo, secondo i Verdi, ha il dovere di affrontare e dare risposte a tali quesiti, senza nascondersi in modo burocratico dietro ad un ordine del giorno del Consiglio comunale, che certamente ha il suo peso, ma che non risolve in alcun modo i problemi di partecipazione dei cittadini e di responsabilità propri del Governo. Mi auguro - e lo spero ancora - che vengano date risposte a queste domande e vorrei concludere chiedendo ancora una volta, un'ennesima volta, al Governo di ripensare questa decisione, proprio in coerenza con quei contenuti e con quel metodo che, almeno per me, sono fondanti per la nostra coalizione dell'Unione.

quel popolo, quei 4 milioni e mezzo di persone andate spontaneamente ad esprimere il proprio parere sul candidato *Premier* di questa maggioranza, di questo che adesso è il Governo del Paese. Siamo la parte che si è sempre mobilitata spontaneamente e volontariamente. Siamo la parte che sente che i propri cittadini non sono stati interpellati e sono stati esonerati dal prendere una posizione di responsabilità. la maggior parte delle affermazioni che ha sentito fare da questa parte. Di là si è esibito un museo delle cere che ha ricordato il passato, un passato che le ultime elezioni americane hanno radicalmente trasformato. Siamo di fronte ad un paesaggio completamente diverso. Chi ama l'America sa che è cambiata, è vicino a questa America cambiata e vuole ragionare insieme con questa America profondamente diversa, rappresentata adesso dalla Camera e dal Senato e in particolare dalla Commissione esteri del Senato americano che ha votato una mozione, a firma Joseph Wien, Ted Kennedy, John Cherry ed altri, nella quale chiede al Presidente degli Stati Uniti di fermare al momento le attività e gli insediamenti militari mentre pende la discussione sul destino della guerra in Iraq. Sono fatti accaduti, fatti di cui sarebbe bene tener conto in una Aula come questa. Ma è lo spirito di profonda abitudine alla vita americana che mi induce a ricordarle un paio di situazioni. Se noi fossimo il Senato americano, adesso ciascuno di noi avrebbe di fronte la mappa delle cose effettive che dovrebbero essere costruite. Vedremmo i passaggi, i luoghi e i punti e non staremmo a discutere su una cosa che non è in discussione, l'amicizia con gli Stati Uniti. Non saremmo a discutere sulle bandiere che non sono in discussione; non staremmo a discutere in particolare, mentre parliamo della città di Vicenza, dell'assetto mondiale internazionale se non per le legittime aspirazioni di pace che motivano appassionatamente questa parte dell'Aula e della maggioranza che rappresenta. Ma sapremmo di più e non sappiamo.

di lavori che i senatori e i deputati avrebbero dovuto approvare. Stiamo discutendo sul vuoto. Sentiamo dai cittadini di Vicenza di tutte le parti lanciare allarmi molto grandi per l'invasione della loro città, che non sono affatto antiamericani perché le colate di cemento non sono né americane né antiamericane, ma sono colate di cemento quando accadono. Le domando, signor Ministro, perché anche lei conosce bene la realtà americana

Qui poi c'è un equivoco: da una parte, si prendono decisioni generali che riguardano il mondo e i cittadini di Vicenza se ne devono fare carico; dall'altra, si dà al sindaco di Vicenza il compito di parlare con i suoi cittadini. Manca un passaggio, signor Ministro,

per città, si sedeva con i cittadini che volevano presentarsi nell'aula magna della scuola più grande o dell'università del centro e discuteva, ascoltando le obiezioni e rispondendo da Presidente degli Stati Uniti? È quel modello americano che abbiamo in mente quando diciamo che non ci convince il modo in cui è stata condotta tale questione. La preghiamo di farsi portatore del disagio, del senso di solitudine e della passione con cui stiamo cercando di impedire che davvero, nel caos e nel malinteso, sorgano sentimenti antiamericani che nessuno di noi vuole e di cui anzi siamo gli antagonisti.

Signor Presidente, signor Ministro, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, ci penserei bene prima di procedere all'allargamento della base americana a Vicenza. Le basi militari Usa nel mondo sono oltre 850, in Europa 499: in otto di esse sono custodite 480 testate nucleari.

Conosciamo le spese militari degli Usa nel nostro Paese, nonché le spese sostenute dallo Stato italiano, non grazie a dichiarazioni dei nostri Governi (noi sappiamo tacere!), ma dall'ultimo rapporto ufficiale reso dal Dipartimento della difesa degli Stati Uniti. Il contributo annuale alla difesa comune versato dall'Italia agli USA per le spese di stazionamento delle Forze armate americane è pari a 366 milioni di dollari,

Quello che le imprese del Nord-Est e del Meridione chiedono disperatamente da anni, gli Usa lo incassano in silenzio già da tempo. «La base si può fare, ma senza carri armati», ha dichiarato il ministro Parisi il 28 settembre 2006. E che cosa ci facciamo, signor Ministro, in quelle basi, coltivazioni biologiche? Che accadrà oltre il filo spinato, nel territorio americano? I giornali dicono che Vicenza avrà in grembo un'unità d'assalto con caratteristiche esclusivamente offensive, ospiterà unità atte a garantire il massimo della potenza nel minimo tempo per tutte le operazioni in Medio Oriente e nei cosiddetti Stati canaglia. Quella di Vicenza sarà la base militare più grande d'Europa; da qui partiranno le forze d'azione per l'Iraq e l'Afghanistan e ogni altra guerra mediorientale per esportare «un cimitero di pace e democrazia» e importare petrolio, in cambio dei quotidiani massacri. In Iraq c'è la guerra che ha mietuto ad oggi oltre 55.000 vittime civili. Il nostro Governo si occupa di moratoria internazionale sulla pena di morte, ma non fa caso che dal Veneto partirà un'armata di distruzione. Ripudiamo la guerra, ma offriamo i nostri territori perché gli altri la facciano! Ma che garbata forma di ipocrisia! Gli Stati ospitanti basi americane, noi tra questi, paghiamo il 41 per cento dei costi. L'impatto del Dal Molin sarebbe di consumi idrici pari a 30.000 abitanti vicentini, gas naturali pari a 5.500 abitanti, energia elettrica pari a 26.000 abitanti. È questo il vostro modo di ripudiare la guerra, com'è scritto nella nostra Costituzione? Dove sono i segni di rottura con il passato? Quali decisioni ha preso questo Governo per imprimere un vero cambiamento, un'inversione di rotta? No, ci spiace, ma non ci stiamo. Mi dispiace dirlo, ma il presidente Prodi ha sbagliato, ha commesso un errore: ha deciso autonomamente, senza neppure consultarsi con il suo Esecutivo, di fare allargare questa base. Al termine della Conferenza stampa gli è poi sfuggito un momento di sincerità, quando ha commentato: «Certo che costruire un aeroporto militare proprio nel centro di una città è un pochino insensato!». Com'è che ha cambiato idea, signor Presidente, arrivando a dichiarare, senza timore del ridicolo, che non si tratta di un problema politico, di una questione meramente urbanistica, che lei non può risolvere perché non è il sindaco di Vicenza. La città palladiana del teatro Olimpico rischia di diventare una Caporetto di questo Governo. Chiediamo, pretendiamo, esigiamo, che il nostro Primo Ministro ascolti i diretti interessati prima di passare all'azione e si consulti anche con noi per decisioni così gravi dal momento che l'Italia è una Repubblica parlamentare. Caro Presidente, l'unica via di uscita, mi dia retta - e sarebbe la prima volta che accade nella storia del mondo - è riconoscere di aver commesso un errore. un atto di umiltà. Sarebbe un gesto straordinario, degno di un *leader* saggio che ascolta la sua gente; un gesto che le farebbe riguadagnare, di colpo, la fiducia che dal giorno dell'insediamento del Governo ad oggi - ad oggi - come dicono i sondaggi - si è parzialmente incrinata. Credo che ne parlerebbero con ammirazione tutti i giornali del mondo. Noi cittadini italiani vogliamo la pace non come alternativa alla guerra, ma come valore assoluto e insostituibile, e la potremo perseguire solo allontanando dal territorio italiano chi la minaccia ogni giorno. Per quanto esposto, dichiaro il voto contrario alle mozioni dell'opposizione.

finestra") *(Ulivo)*. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi,premessa necessaria a questo mio breve intervento sull'ampliamento della zona militare americana a Vicenza è l'esigenza di sottolineare alcuni punti critici che, mi auguro, saranno approfonditi nelle sedi parlamentari, nei tempi più brevi possibili, trovando spazi di confronto anche prima della definizione finale dei programmi di allargamento della base USA. Dopo settimane di forti contrasti e diverse posizioni nell'opinione pubblica, in particolare alimentate dalle proteste della cittadinanza vicentina che, a mio avviso, ha esternato legittimamente la propria disapprovazione verso una decisione non partecipata e completamente condivisa dalla comunità locale poiché ritenuta irrispettosa dei vincoli urbanistici, ambientali ed architettonici, è fondamentale ricordare che sul raddoppio della base americana a Vicenza il Governo Prodi ha compiuto una scelta in base agli impegni già presi dal precedente Governo e al via libera del Comune di Vicenza che, infatti, aveva già concesso l'autorizzazione. Se negare l'ampliamento adesso sarebbe «un arbitrio e un atto di ostilità» nei confronti degli Stati Uniti, è quindi necessario considerare la scelta già compiuta. Condivido allora la proposta del ministro degli affari esteri D'Alema di rivedere il progetto, garantendo, pertanto, un minore impatto sulla città. Sono confortata dall'impegno del ministro della difesa, Parisi, che assicura una vigilanza affinché tutte le opere programmate per Vicenza siano rispettose delle esigenze rappresentate dalle comunità locali, con particolare riferimento all'impatto sull'ambiente, sul tessuto sociale, sulla viabilità e sulla rete dei servizi. Mi auguro possano nascere da questi impegni annunciati le nuove linee per la nostra politica, senza contrapposizioni e spaccature ideologiche, che poco fanno se non provocare uno scontro fondato su posizioni pregiudizialmente a favore o contro, fino all'identificazione delle basi alleate con il potere militare degli Stati Uniti. Tutto questo senza neppure, o solo lontanamente, sfiorare il cuore del problema da cui dovrebbe scaturire un dibattito serio sull'utilità, sui costi e sulle funzioni delle basi militari relativamente al principio di tutela dell'interesse nazionale, al principio di sovranità e sul piano della legalità internazionale a quello di reciprocità. Reciprocità che caratterizza i nostri accordi bilaterali con gli Stati Uniti in materia di utilizzo delle basi relativamente agli impieghi operativi. È rispettata, però, la condizione di reciprocità se non sono neppure prese in considerazione proposte di siti alternativi alla base di Vicenza? C'è reciprocità se una decisione viene subita e non condivisa? Sono davanti a tutti noi le indubbie responsabilità del Governo Berlusconi e del Comune di Vicenza, che sono state purtroppo determinanti nella pessima gestione dell'ampliamento della base e, soprattutto, nella totale mancanza di coinvolgimento della società civile; ma il problema è anche più ampio. Ritengo che se due Stati sovrani non sono in grado di confrontarsi e di «trattare», nel senso più politico del termine, su decisioni da assumere che riguardano per giunta la collettività, allora siamo in evidente stato di assenza di «reciprocità». Allora l'interesse nazionale di uno dei due Stati è superiore all'altro e, ignorando la presenza di accordi segreti, ritengo che questo sia profondamente inaccettabile, come sono inaccettabili tutte quelle forme di velati o palesi *aut aut*. Esiste una sovranità ed è quella che ogni Stato esercita sul proprio territorio. Esiste una reciprocità ad esempio in altri campi, come nella cooperazione giudiziaria in materia penale. Viene sempre rispettata da entrambe le parti? Difficile rispondere positivamente quando sono ben visibili tutte le gravi incongruenze che, attraverso le più varie misure adottate dalle istituzioni in questi anni, creano enormi difficoltà sotto due profili specifici: quello delle garanzie procedurali nei procedimenti penali e quello del necessario bilanciamento tra attività di prevenzione e repressione del terrorismo e salvaguardia dei diritti umani fondamentali. È necessaria quindi una reciprocità se si vuole applicare una reale cooperazione, perché siamo alleati non sudditi. Cosa ci può essere di più reciproco di un'alleanza? In questa storica alleanza con gli Stati Uniti noi crediamo e riteniamo che per renderla ancora più solida vada maggiormente implementato il reciproco rispetto delle due parti. Come difendere questo principio di reciprocità relativamente alla decisione di ampliare la base di Vicenza? Tenendo ben distinti i giudizi sulle scelte della nostra politica estera e di difesa che, già da questi primi mesi, stanno trovando segnali forti di un nuovo segno politico. È rilevante concentrare la nostra attenzione sui programmi operativi e quindi sul necessario sforzo per individuare quelle misure capaci di limitare al minimo i danni per la città di Vicenza.

Lascio a voi giudicare se questa è una rappresentazione corretta della mia personale maniera di pormi. Ho già detto personalmente al sindaco che le sue argomentazioni mi sembrano formalisticamente corrette, ma se la popolazione protesta vuol dire che c'è un problema politico del tutto aperto. Naturalmente, se manca la seconda parte la prima assume tutto un altro significato. Non sono abituata ad occuparmi molto delle cose che mi riguardano personalmente e quindi desidero andare avanti

attraverso dichiarazioni - mi perdoni il Ministro non presente - alquanto burocratiche viene fuori un protagonismo della popolazione che ha i caratteri, per la prima volta dopo un po' di tempo, dell'affermazione sostanziale della sovranità popolare. È questo il caso di Vicenza, non sono forze politiche che insufflano qua o là, come è risultato chiaramente anche negli interventi precedenti, specialmente quello della senatrice Valpiana. E' là sovranità popolare che si esprime nella sua nativa forza: la base dello Stato. Su questo nessuno può permettersi né sottovalutazioni né irrisioni.

orientamenti che ci consentirebbero di agire, quando Jimmy Carter, la manifestazione di Washington mostrano un mutamento negli equilibri politici degli Stati Uniti, quando si rimette in moto con fatica la costruzione dell'Europa e quindi le relazioni tra le grandi potenze del mondo vengono ridiscusse, torna alla base la politica, la sovranità popolare fondamento della sovranità nazionale. È questa la grande offesa che Vicenza ci manda a dire, e manda a dire per sé ma per tutti, perché la sovranità popolare, quando si esprime in un punto, riecheggia in tutta la popolazione, in tutta la cittadinanza. Per questo ci sarà una manifestazione nazionale a Vicenza: perché questo è il valore politico della questione e se non lo cogliamo, andando anche oltre le nostre incapacità di capire e le nostre difficoltà, credo che non rispondiamo a questa grande istanza e non teniamo conto, perciò,

«contro di me sconfitto», perché si fece carico della sconfitta, che pure non aveva provocato, né subito - «tranne la vostra personale cortesia». Gli rispose Churchill, che pure non era un tipo tanto dolce e che tuttavia riconobbe che in quel momento De Gasperi rappresentava una sovranità popolare che non aveva nemmeno ancora potuto esprimersi in modo formale, che raccoglieva la Resistenza, Cefalonia, i 750.000 internati militari italiani, il Corpo italiano di liberazione, che era risalito insieme all'esercito americano e agli altri; non c'era niente di formalizzato, ma c'era sostanzialmente la sovranità nazionale e la sovranità popolare. Questa si ripresenta ad una svolta della storia e se non ce ne rendiamo conto, secondo me, siamo inferiori al ruolo che rappresentiamo: cerchiamo di evitarlo. Signor

alla mia interrogazione. Un Paese serio mantiene gli impegni e non si può impedire ad un Governo l'assunzione doverosa di responsabilità. Dobbiamo tenere fede ad un rapporto tradizionale di alleanza ed al principio della continuità istituzionale con gli impegni che i Governi si assumono. Come il ministro Parisi ci ha riferito stamane, la questione dell'ampliamento della base non è un novità per il Governo italiano: è infatti nell'ottobre 2004 che giunge al Governo la prima richiesta orientativa per l'autorizzazione ad utilizzare le infrastrutture e le e le aree dell'aeroporto Dal Molin e il Governo italiano allora manifestò il proprio parere favorevole e d'interesse. Nell'anno successivo al perfezionamento delle richieste americane, sono stati dati pareri tecnici favorevoli ed è sempre stata dichiarata la disponibilità massima delle autorità politiche della difesa italiana. L'atteggiamento ostile di alcuni colleghi oggi porta solo a mostrare l'Italia come un Paese pieno di contraddizioni e ambiguità, che non ricorda il suo passato e il suo contributo alla politica estera dell'Alleanza atlantica. Da cittadino veneto, capisco realmente le preoccupazioni manifestate all'interno della comunità locale, ma vorrei evidenziare che, su richiesta espressa del Governo, c'è stato un pronunciamento esplicito del Consiglio comunale, arrivato lo scorso 26 ottobre, su un ordine del giorno che condiziona il sì all'ampliamento al rispetto di cinque condizioni: assenza di voli militari connessi con l'attività operativa del reparto USA; esonero dell'amministrazione comunale da qualsiasi spesa per la realizzazione anche delle infrastrutture viarie; assenza di impatti negativi sull'attività dell'aeroporto civile; salvaguardia o trasferimento dell'attività sportiva oggi esistente nell'area; impegno dell'amministrazione americana ad utilizzare risorsa professionali locali. Quindi, mi pare chiaro che alla base di questa decisione ci sia il rispetto delle comunità locali e la considerazione dell'impatto sul tessuto sociale stesso. È fuori da ogni dubbio che con il sì all'allargamento della base si andranno a sviluppare nuovi scenari che impongono una necessaria valutazione da affrontare in via preliminare. L'aumento della popolazione residente, il congestionamento della rete viabilistica, così come l'aggiornamento della funzione commerciale e turistica sono alcuni temi derivanti dal progetto Dal Molin che vanno considerati e chiaramente risolti. Ma sono sicuro che le autonomie locali troveranno le soluzioni adatte per armonizzare le politiche di sviluppo con le istanze delle categorie interessate. E non vedo come non si possano coniugare le esigenze dei cittadini con un'opportunità di vantaggio economico e di immagine per l'Italia e per il Veneto. Pensare di essere sottomessi ad un atto di colonizzazione è un atteggiamento retrogrado e di chiusura che non giova allo sviluppo dell'Italia che oggi, soprattutto, ha la necessità di dimostrare la reale volontà di cambiamento e l'apertura alla modernità non con parole ma con pragmaticità e chiarezza. La nostra politica estera non può farsi condizionare dalla demagogia antiamericana. Il rapporto dell'Italia con la NATO ed un rapporto particolare con gli Stati Uniti serve a consolidare la pace, la stabilità e la difesa dei diritti. Ricordiamoci che il sì all'ampliamento della base, oltre ad essere un successo politico per l'Italia, porterà nuovi posti di lavoro e nuova ricchezza ai cittadini, mentre la chiusura della "Ederle" toglierebbe lavoro a circa 750 persone, alle rispettive famiglie e metterebbe in difficoltà molte aziende con ricadute negative sull'intera comunità. L'economia veneta e italiana non può permettersi di subire questa retrocessione. Alle reazioni di chi ha dichiarato che dalla base di Vicenza possono partire azioni di guerra, ricordo (come sottolineato nella mozione di alcuni miei colleghi), che nel marzo 2003 una deliberazione del Consiglio Supremo di Difesa, nel proclamare la condizione di non belligeranza della Repubblica italiana nei confronti, ad esempio, dell'Iraq precluse esplicitamente al Governo degli Stati Uniti di avvalersi delle proprie basi sul territorio nazionale italiano per attaccare direttamente bersagli siti nel territorio iracheno, inclusa quella di Vicenza. A conclusione del mio intervento chiedo ai colleghi di rendersi scevri da ogni sovrastruttura mentale e analizzare il problema in termini di opportunità per il nostro Paese, per il Veneto e per la città di Vicenza.

la votazione odierna è particolarmente delicata poiché il vero nodo della questione non è l'opportunità o meno dell'ampliamento della base USA di Vicenza, bensì la modalità dell'*iter* attuato e attuale. Personalmente non intendo sindacare le linee di politica estera seguite, sia dal precedente Governo che da quello attuale, riguardo l'inclinazione filoamericana con cui preserviamo un vincolo di alleanza e di amicizia decennale. Tuttavia, nella fattispecie credo necessario procedere in un'ottica di cauto equilibrio. Colleghi, vi esorto a riflettere sulla vicenda da un'angolazione diversa, accantonando l'amicizia atlantica, che ci lega agli alleati americani, per focalizzare la questione nel merito e alla luce delle istanze locali. Siamo certi che per i vicentini l'ampliamento corrisponde a sviluppo economico e incremento occupazionale, ma ciò è propedeutico all'impatto ambientale, urbanistico e sociale; da questa ottica, pretendere un giudizio di fattibilità che coinvolga i soggetti interessati è regola di democrazia. È troppo facile dire sì quando non si è direttamente compromessi; il nostro sì invece sarà subordinato a un provvidenziale confronto che dia voce alla posizione di Vicenza. Quindi, al monito dei colleghi che argomentano sull'affidabilità nei confronti degli USA per richiamare il Governo al rispetto dei patti, con franchezza ribatto che un Paese, ancor prima di onorare gli accordi, ha obblighi di rispetto democratico verso i suoi cittadini. Pertanto, è d'uopo porre la questione avendo presente sia un coinvolgimento da parte delle popolazioni locali che la problematica procedurale, giacché, trattandosi di accordi internazionali, il dibattito parlamentare che ne approvi natura e condizioni è presupposto vincolante. Così però non è stato. Infatti, nella precedente legislatura il Parlamento non ha avuto la possibilità di valutare preventivamente il caso, dando il giusto orientamento al Governo, e ciò ha determinato un grave

a nome dei Popolari-Udeur, manifesto il mio voto contrario alle mozioni presentate dall'opposizione, certo che il Governo opererà concretamente, nel più breve tempo possibile, tenendo presenti le esigenze della comunità vicentina. Devo dire che avrei preferito che in quest'Aula la maggioranza avesse presentato una propria posizione chiara. Ciò non è accaduto e spero che succederà nei prossimi minuti.

Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghe e colleghi, la decisione del Governo di autorizzare l'ampliamento della zona militare americana di Vicenza ha aperto un dibattito tra le forze politiche e ha suscitato contrasti, anche aspri, tra i cittadini vicentini e, più in generale, nell'opinione pubblica. Alla base di queste contrapposizioni, vi sono, da un lato, ragioni di politica estera e di difesa, tese a mettere in discussione una scelta dell'Amministrazione degli Stati Uniti d'America, che, nell'ambito di una strategia di riduzione e di ricollocazione delle proprie Forze armate in Europa, punta al potenziamento delle capacità della brigata di stanza a Vicenza. Dall'altro, vi sono ragioni più immediate, poste in primo luogo dai cittadini di Vicenza, che riguardano gli effetti possibili dell'impatto ambientale derivante dal raddoppio della base militare, che si trova peraltro nel cuore dei quartieri residenziali della città. Signor Presidente, colleghi, è per noi chiaro che vanno nettamente tenuti distinti i giudizi sulle scelte di politica estera e di difesa che il Governo ha legittimamente adottato, nel rispetto degli accordi di collaborazione bilaterale politico-militare tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, da quelli sulle posizioni di quanti paventano rischi seri per le conseguenze dell'impatto ambientale sulla città Vicenza. Per quanto ci riguarda, non possiamo non preoccuparci delle riserve e dei dubbi espressi da più parti della comunità vicentina. Tali dubbi e riserve esprimono non un sentimento antiamericano, ma la paura di un impatto rilevante sulle condizioni di vita della comunità vicentina. Noi abbiamo il dovere di dialogare con questa nostra comunità. Come ha ricordato la senatrice Valpiana, anche in sede parlamentare, qui al Senato, avanzammo la richiesta di un pronunciamento più esteso da parte dei cittadini, senza pregiudizialmente pronunciarci noi contro o a favore dell'ipotesi di "Ederle 2", ma chiedendo che la popolazione vicentina, prima del 26 ottobre 2006, data nella quale il consiglio comunale avrebbe assunto una decisione in proposito, avesse l'opportunità di pronunciarsi. Altresì abbiamo il dovere di tutelare l'affidabilità delle relazioni e degli impegni internazionali che il nostro Paese ha assunto, tanto più quando questi attengono a strategiche alleanze politiche e ai conseguenti patti militari;

o quella maggioranza politica e che non possono essere delegati a decisioni di singole, per quanto importanti, realtà territoriali. Dunque, il Governo ha risposto positivamente alla richiesta di ampliamento della base avanzata nel 2004 dal nostro principale alleato e Paese amico, gli Stati Uniti, perché tale richiesta è compatibile con gli accordi assunti in coerenza con le linee della politica estera e di difesa del nostro Paese. Peraltro, anche i deliberati della rappresentanza istituzionale locale e segnatamente del Consiglio comunale di Vicenza si sono espressi nello stesso senso con l'approvazione di un ordine del giorno del 26 ottobre 2006, che dà parere favorevole all'accoglimento nel territorio comunale di Vicenza della 173a Brigata aviotrasportata degli Stati Uniti. L'auspicato, in sede parlamentare, come detto, e dallo stesso Governo diretto pronunciamento dei cittadini non vi è stato, perché può deciderlo solo il Comune; non certo l'Assemblea, non certo il Governo per esso. Tuttavia - e questo non può che essere apprezzato - il Governo si è posto esso il problema della sostituibilità territoriale e di misure per ridurre l'impatto della "Ederle 2" coerentemente con un approccio nuovo in materia di di strutture militari, cui faceva riferimento la senatrice Donati nel suo intervento. A questo proposito, vorrei ricordare che si sta procedendo a riunioni bilaterali, dedicate alla problematiche delle singole Regioni; in particolare, si è iniziato con la Sardegna ed il Friuli-Venezia Giulia a formare i primi elementi di beni militari dismissibili. Nella stessa linea di condotta vanno riportate le azioni che hanno definito la cessione di Palazzo Barberini, l'iniziativa relativa alla cessione delle frequenze WiMAX, che per territori dell'interno del territorio nazionale, laddove il segnale del GPS non è possibile sia utilizzato, è di fondamentale importanza per le comunicazioni, nonché il rilascio da parte della Marina militare statunitense della base militare della Maddalena. Il Governo, quindi, non ha cambiato idea rispetto ai contenuti delle linee indicate nel programma. Voglio anche ricordare che nella finanziaria, poche settimane fa approvata, si prevede un programma di dismissione dei beni immobili in uso alla difesa per un valore di quattro miliardi di euro in due anni. Tornando al problema specifico al nostro esame, in ogni caso ritengo sarebbe doverosa una corretta informazione innanzitutto sulla assoluta insussistenza di progetti che riguardino l'utilizzo militare dell'aeroporto di Vicenza, che resterà all'aviazione civile, ed inoltre che nella "Ederle 2" non sono previste attività belliche di diretta pertinenza della base. Dunque, gli Stati Uniti vi organizzano e concentrano le forze in termini di comando e di logistica. Le scelte di politica estera non possono e non debbono essere ridotte a semplici autorizzazioni amministrative, né allo stesso tempo, però, possono essere elemento di ambiguità ed equivoci tanto più quando da esse dovessero derivare lesioni alla limpida e robusta lealtà nei confronti dei nostri alleati, ed in questo caso del nostro principale alleato. Negare l'ampliamento ora, dopo gli impegni assunti, equivarrebbe ad un atto ostile. Ecco perché io penso che il Governo abbia correttamente e coerentemente assunto una determinazione ed in tal senso sosteniamo quanto a nome del Governo, per le ragioni e le motivazioni qui portate dal Ministro della difesa,

lunedì scorso sono stato a Vicenza per prendere parte ad una assemblea di comitati di cittadini che si oppongono all'ampliamento dello spazio della base militare statunitense. L'incontro si realizzava in una grande sala all'interno della stupenda chiesa della Santa Corona. Non ho potuto entrare, io e centinaia di altre persone, perché il locale era pieno. Insieme con altri colleghi parlamentari abbiamo proposto di tenere un'assemblea parallela per poter ascoltare le posizioni che i partecipanti desideravano esprimere. Ciò che si fece in piedi al freddo serale nel chiostro della chiesa domenicana e per due ore e mezzo abbiamo ascoltato i reclami indignati di quella parte degli abitanti di Vicenza e dei Comuni di Dueville e Caldogno. Una delle dichiarazioni più frequenti era che non potevano più avere fiducia nei politici istituzionali perché si sentivano traditi dal Governo. Ho promesso che quello che dicevo lì direttamente ai presenti, lo avrei ripetuto in Parlamento e in qualunque altra sede istituzionale. In questo senso approfitto del poco tempo di cui dispongo per fare un riassunto di quello che ho detto a Vicenza e che è stato quanto segue. Ho avuto la fortuna di essere uno dei fondatori del *Forum* sociale mondiale di Porto Alegre nel 2001, che tra l'altro ha terminato un'ulteriore sessione di lavori pochi giorni fa a Nairobi. Là il nostro movimento è nato con una serie di parole d'ordine e di campagne, ma tre pilastri erano e sono basilari: la lotta contro la guerra; la difesa dei beni comuni; la democrazia partecipata. Ed ecco che i diversi comitati vicentini, volenti o nolenti, che lo sappiano oppure no, si sono trasformati in questo momento nell'avanguardia italiana di queste tre rivendicazioni. La base Dal Molin è strategica e non ha niente a che fare con la difesa: la sua funzione è aggredire altri popoli, che non sappiamo neanche quali potranno essere, nell'Est europeo o nel Nord Africa. E' un peso difficile da sopportare per chi possiede un'anima e un cuore. Quella immensa struttura militare sfregia la natura, distrugge i boschi, aggredisce il bacino idrico e annichilisce la meraviglia storica ed architettonica della città e delle ville, dichiarate dall'UNESCO patrimonio dell'umanità. Colpisce quindi, e profondamente, il bene comune dei veneti e di tutta l'umanità. Quella comunità che credeva nella democrazia in questo momento si sente umiliata: come mai si chiede - il Governo che aveva promesso di prendere la strada della pace marcia per la guerra e dice che lo fa perché ci sono dei patti, a dire il vero molto fumosi, con gli USA? E ancora E ancora si domanda: e con noi non esiste nessun patto? Non si discute, non si ha il coraggio di presentarsi fra questi italiani? Caro Presidente,

Presidente, onorevoli colleghi, la vicenda relativa all'allargamento della base militare di Vicenza sta assumendo i contorni di un incredibile giallo, rispetto al quale la popolazione di quella città e di quella Regione ha certamente il diritto di pretendere chiarezza rispetto a comportamenti istituzionali inspiegabili. Comportamenti che se non appartenessero alle esposizioni di autorevoli esponenti del Governo e della politica rischierebbero di apparire realmente ridicoli. considerato che la Commissione difesa, che ho l'onore di presiedere, ha recentemente approfondito l'argomento nell'ambito di una missione cui hanno partecipato senatori di maggioranza e opposizione. Il dato più inquietante è quello relativo alla non conoscenza da parte del presidente del Consiglio Romano Prodi dell'impegno assunto per l'ampliamento della base americana: «Non ne sapevo nulla», dichiara a caldo il presidente Prodi, e io da parlamentare resto allibito, onorevoli colleghi, perché è improbabile che tali intenzioni non siano certificate nell'ambito degli accordi politico‑militari che regolamentano i nostri rapporti con gli alleati. La mia richiesta è quella quindi di conoscere se esistano protocolli militari coperti dal segreto di Stato, dei quali il presidente del Consiglio Prodi abbia preso almeno visione. Lo strumento dell'audizione presso le competenti Commissioni parlamentari dei soggetti detentori della consuetudine di rapporto con le autorità militari statunitensi potrebbe quindi rappresentare un elemento di chiarezza rispetto ad un'operazione verità che questo Parlamento ha il diritto di pretendere. Onorevoli colleghi, non intendo mettere in discussione la ricostruzione del ministro Parisi, tutta legata a documenti epistolari protocollati in data certa, ma credo fermamente che qualcosa in più ne sappiano il direttore del SISMI dell'epoca, il Capo di Stato maggiore della Difesa e perfino il Sindaco di Vicenza che alla Commissione difesa ha raccontato di uno scambio epistolare, definito surreale, atto a respingere il tentativo di lasciar credere che le decisioni sulla base americana da ampliare potessero in qualche modo semplificarsi ad atti amministrativi di pertinenza della politica locale. locale. Onorevoli colleghi, sia chiaro: chi vi parla è convinto che l'ampliamento della base rappresenti un valore aggiunto per Vicenza dal punto di vista della ricaduta economica e che nulla di strategico rappresenti quell'insediamento se non la struttura di permanenza residenziale di ulteriori 1.600 militari in aggiunta a quelli già stanziali.

Signor Presidente, colleghi, il dibattito di oggi e la vicenda di cui ci stiamo occupando dimostrano alcuni aspetti surreali

l'alleanza che, dalla fine della Seconda guerra mondiale, ci lega agli Stati Uniti fosse profondamente radicata nelle coscienze e nelle forze politiche e parlamentari di questo Paese, probabilmente questo dibattito non ci sarebbe stato. Ci saremmo infatti trovati in una situazione in cui, in un normale rapporto di alleanza, l'ampliamento l'ampliamento della base sarebbe stato in sé, senza che si dovessero mobilitare cittadini pro o cittadini contro e senza che questa potesse diventare una questione che mette in qualche modo a repentaglio anche la vita del Governo. In realtà, quello che si dimostra è che nel nostro Paese, nel Parlamento

è elevatissima, rilevantissima e non attinge soltanto ad alcune forze politiche, ma ne attraversa tutto lo spettro. Quest'oggi abbiamo sentito

sorprendenti che provengono non soltanto da settori della sinistra radicale. Il collega Colombo ci accusa di essere il museo delle cere perché saremmo ancorati a vecchie visioni. Voglio solo far notare che che nelle anomalie della democrazia italiana siamo arrivati al punto che, nonostante nella maggioranza di Governo, tra i partiti che la compongono e tra gli esponenti che sono in questo Parlamento e al Governo sia una profonda divisione sulle decisioni, il dibattito parlamentare si deve solo al merito dell'opposizione che ha presentato documenti e che ha chiesto che questa discussione avvenisse. È francamente paradossale che una maggioranza di Governo, che ha fatto del parlamentarismo la sua bandiera fondante e che su questo ha giocato e vinto un *referendum* costituzionale, nel momento in cui ha un problema politico decida di scavalcare il Parlamento e che, se non fosse stato per l'opposizione, in Parlamento non si sarebbe discusso. Dico ai colleghi che si sono espressi contro le decisioni del Governo che il loro attaccamento al potere è superiore alle loro convinzioni, tanto che non hanno provocato loro questo dibattito, ma l'abbiamo fatto noi. Voglio ora tornare al tema di fondo, all'antiamericanismo che pervade oggi molti colleghi. La collega Calipari

americana a Vicenza non si sarebbe dovuta fare. Quindi, la posizione vera della collega Calipari non è di favore all'ampliamento della base, ma di contrarietà,

questa è coniglieria istituzionale elevata a posizione politica per mediare con coloro, come alcuni colleghi di Rifondazione (non tutti, perché il collega Nieddu ha detto cose diverse dalla collega Menapace), che sono ancorati, loro sì museo delle cere, caro Colombo, loro sì antiquariato o anticaglia della peggiore corrività con le dittature dello scorso secolo! Noi abbiamo vissuto, caro Colombo, in una situazione nella quale il maggior partito di opposizione era al soldo del nemico storico di questo Paese! *(Applausi dai Gruppi FI e AN)*. E solo la presenza americana e la politica degli Stati Uniti ha garantito che tu, collega Colombo, sieda in questo Parlamento e non in una *duma*.

La verità è che il Governo non ha una maggioranza in politica internazionale o, meglio, non ha una politica internazionale *tout* *court*. Il Governo dovrebbe, se fossimo una democrazia seria e matura, misurarsi in questo Parlamento con una decisione ai voti non su mozioni dell'opposizione, ma sulla decisione stessa di consentire l'ampliamento della base di Vicenza. Avrebbero dovuto avere tale coraggio, se ce l'avessero (ma chi

che dobbiamo rompere il più possibile questa alleanza, abbandonando l'Afghanistan, dopo aver abbandonato l'Iraq, e magari abbandonando altre cose. Ma c'è, forse, nella storia recente un punto che mi preme sottolineare. Quando la sinistra si è trovata ad avere responsabilità dirette di Governo ed era Presidente del Consiglio l'attuale ministro degli affari esteri Massimo D'Alema, dalle basi americane in Italia sono partiti aerei che hanno bombardato la Serbia. All'epoca non ero in Parlamento, signor Presidente, ma ho plaudito a quella decisione e al senso di responsabilità internazionale ed istituzionale e al rigore della mia parte politica, che sostenne quella decisione di Governo con il voto in Parlamento, non cedendo alla facile tentazione di usare la politica internazionale di un Paese, che ancora mi risulta essere tra le sette potenze industriali del mondo, industriali del mondo, per far cadere un Governo sulle sue contraddizioni, mettendo in gioco la credibilità internazionale del Paese. Ebbene, oggi il Governo rivela la sua codardia istituzionale, la codardia di alcuni suoi esponenti, con la mancanza del coraggio di riconoscere

È la piazza di Vicenza - ci ha detto la collega Menapace - che deve prevalere rispetto alle decisioni del Parlamento. Hai ragione, collega Menapace, perché, grazie alla tua maggioranza, al tuo Governo e al Presidente del Consiglio che tu sostieni,

anche rispetto ai vostri proclami pacifisti, non interventisti, terzomondisti. Essi fanno parte non del museo delle cere, ma del magazzino

che ha sostenuto l'ingresso del Venezuela di Chavez nel Consiglio di sicurezza dell'ONU *(Applausi del senatore Amato).* È una vergogna per un cittadino italiano che crede nei valori fondanti della Repubblica essere governato da questa maggioranza e da questo Governo.

colleghe e colleghi senatori, il nostro dibattito verte su un tema che può apparire relativo da un punto di vista politico generale, in quanto si tratta di dare seguito ad impegni internazionali che il nostro Paese ha assunto a livello non solo europeo, ma anche all'interno dell'Alleanza atlantica e delle Nazioni Unite. Credo, cari colleghi, che dobbiamo essere onesti con noi stessi, capendo fino in fondo che qui non si tratta soltanto di decidere se allargare una base militare. Mi sembra che il contenuto del nostro dibattito, che nessuno vuole far apparire così com'è, nella sua piena autorevolezza politica, sia di tutt'altra natura. Oggi discutiamo della politica estera del nostro Paese e ci chiediamo se la maggioranza che governa in questo momento l'Italia sia in grado di esprimere una politica estera e un supporto agli accordi internazionali che l'Italia stessa ha assunto, anche in passato. Mi sembra che questa sia la ragione per la quale abbiamo riscontrato - non solo in questa vicenda ma anche in altre occasioni - le grandi difficoltà del Governo ad assumere decisioni in politica estera. Abbiamo visto il Ministro degli affari esteri impegnato in diverse occasioni e smentito quotidianamente dai suoi vice Ministri o dai membri della sua maggioranza e del Governo.

(in considerazione anche del fatto che in questo biennio siamo impegnati in Consiglio di sicurezza) ci fanno capire sempre di più che l'Italia deve mantenere il prestigio internazionale che la storia e la politica il prestigio internazionale che la storia e la politica di questi ultimi vent'anni hanno affidato al nostro Paese - non solo nel Mediterraneo, ma anche in Europa, per la costruzione dell'Europa per le grandi intuizioni della politica italiana e che non può essere svenduto per un fatto ideologico o per questioni interne ad una maggioranza. Qui c'è in gioco il futuro delle nuove generazioni di italiani e di europei.

negli ultimi sei mesi, stiamo facendo passi indietro e stiamo perdendo credibilità internazionale. La chiarezza, cari colleghi della maggioranza e del Governo, è uno dei presupposti importanti per rendere dignitoso un Paese. Se ci sono delle divergenze nel Governo, se ci sono delle divergenze nella maggioranza, è bene esprimerle qui, ufficialmente, senza nascondersi dietro a delle mozioni che dicono tutto e il contrario di tutto e che hanno lo scopo di dire ai militanti della sinistra estrema: «Stiamo lavorando per evitare che questo avvenga». Nel frattempo, però, si fa un occhiolino al Governo perché non vuole perdere il potere, perché tutti sanno che una divisione in politica estera nel nostro Paese, in questa maggioranza, in questo Governo significherebbe la sua stessa fine. allora che le coscienze possono essere appagate soltanto con la chiarezza. Parlate in Parlamento, in questa Camera, colleghi dell'opposizione, come bene ha fatto il senatore Nieddu, il quale ha espresso con chiarezza la sua posizione, la vocazione di Governo anche nel suo intervento, rispettando i patti internazionali, rivolgendosi anche ai suoi militanti di Rifondazione Comunista, della sinistra. della sinistra. Quelli che dissentono da questa posizione debbono dirlo e non debbono nascondersi dietro un impegno più lato, più generale di mantenere la coalizione di Governo.

Parisi ha dichiarato chiaramente che procederà anche in questa direzione e noi daremo tutto il nostro appoggio. Come lei ben sa, Presidente, e concludo, l'UDC e l'opposizione in generale hanno dato sempre in materia di politica estera il segnale, non nel Parlamento, non nella politica interna ma all'esterno, della garanzia della continuità degli impegni internazionali. E' tale vocazione che in questa opposizione momentanea di oggi dobbiamo portare avanti. È per questa convinzione che siamo forza di Governo. Siamo forza di Governo perché siamo consapevoli che la nostra forza deriva dalla storia, dalla conferma dei patti assunti, perché soltanto con la loro conferma un grande Paese come l'Italia può fare passi avanti.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, la questione che esaminiamo oggi mi pare debba essere oggetto di due tipi di approccio: l'uno che concerne la città di Vicenza, i suoi amministratori e i suoi abitanti; l'altro, invece, che consideri più generalmente il significato dell'ampliamento della presenza militare americana sul territorio italiano. Sono il rappresentante di una Regione fortemente attaccata alle sue peculiarità e alla sua autonomia e prima ancora un convinto assertore dei valori del federalismo. Mi pare perciò doveroso richiamare l'attenzione sulla necessità di essere estremamente attenti alla volontà e alle esigenze della popolazione vicentina. Perché ciò sia possibile, mi permetto di sottolineare quanto sia necessario che essa sia perfettamente informata di tutte le implicazioni che la costruzione della nuova base americana comporterebbe. Quale che sia l'esito del procedimento in corso, occorre comunque che esso sia improntato alla massima trasparenza, a maggior ragione quando si parla di insediamenti che, per la loro stessa natura, comportano anche una forte carica simbolica e che possono essere percepiti come rischi. Si dirà che a sottomettere qualunque realizzazione alla volontà della popolazione locale nulla sarà poi effettivamente realizzato, ma non è la mia opinione. Credo e mi auguro che le autorità comunali, in particolare il Consiglio comunale e il Sindaco di Vicenza, abbiano veramente esercitato con senso di responsabilità le loro funzioni di rappresentanza degli abitanti della città di Vicenza, che sappiano valutare rischi e opportunità ed abbiano preso senz'altro una decisione ponderata. Sono convinto che proprio la poca chiarezza del processo decisionale che talvolta circonda queste scelte sia in realtà un motivo di troppi frequenti rifiuti opposti a misure invece necessarie, dai rigassificatori alla TAV: è lungo l'elenco di opere che vengono viste con sospetto proprio perché mal presentate. Informazione corretta e coinvolgimento di tutti gli attori istituzionali nella scelta mi paiono, quindi, la migliore garanzia di successo nella modernizzazione del Paese che passa certo attraverso una chiara definizione della sua struttura militare e dei suoi impegni internazionali. Occorre valutare bene le ragioni dell'ampliamento della base militare di Vicenza, occorre prendere in considerazione le legittime preoccupazioni della popolazione cittadina, alla quale deve essere presentato in modo chiaro il progetto di ampliamento ed il suo impatto sul territorio, sul tessuto socio-economico della città, considerando anche i Comuni vicini e le conseguenze positive e negative che ne possono derivare. Il Parlamento deve conoscere bene le ragioni di questo allargamento - oggi il Ministro ha illustrato, con dovizia di particolari, tutto questo questo processo - e, soprattutto, deve sapere quali sono le finalità della base e quale sarà l'utilizzo di un contingente militare così importante. La decisione finale deve tener conto degli impegni italiani, dell'amicizia e dei rapporti bilaterali con gli Stati Uniti, nel rispetto delle alleanze tradizionali del nostro Paese, anche tener conto dell'evoluzione degli interessi e delle posizioni dell'Italia e dell'Europa allargata nei nuovi rapporti e nei nuovi equilibri politici. Una presenza militare così importante deve essere garanzia per la pace, senza coinvolgerci in avventure di cui magari poco conosciamo, che magari non condividiamo e che potrebbero anche rappresentare dei rischi per la pace nel mondo.

sinistra radicale, si è lasciato andare ad una di quelle affermazioni che lasciano il segno ed inchiodano l'interlocutore alle sue inevase responsabilità verso il Paese. «Il problema» - ha detto - «non è il disaccordo di qualcuno con una particolare scelta del Governo, quanto il fatto che manca ancora una cultura della difesa e della sicurezza e ciò impedisce il dialogo con coloro che scendono in piazza e con i parlamentari dissidenti». A parte il fatto che parlare di dialogo mi sembra fuori luogo - in quanto abbiamo chiesto almeno una decina di volte un incontro con il Ministro - condivido pienamente le che tuttavia farebbe bene a riferire a se stesso. Il dato più grave, infatti, che trapela dalle scelte del Governo sulla base di Vicenza, e sulle questioni delle servitù militari in generale, è proprio la sconcertante mancanza di attenzione per la difesa del territorio, delle comunità che lì vivono dei beni comuni che vi sono presenti, così come non vi è traccia di politiche finalizzate alla reale sicurezza dei cittadini, alla tutela della loro salute e dei loro interessi primari. È una questione di cultura, in effetti, a determinare questa latitanza: per i Governi che si sono avvicendati alla guida del Paese dal secondo dopoguerra in poi, la sicurezza è sempre stata sinonimo di militarizzazione e controllo. Purtroppo, anche il Governo attuale non si sottrae alla regola, con l'aggravante, però, che nel programma con il quale la coalizione di centro-sinistra si è presentata al Paese si affermava, seppur timidamente, di voler invertire la rotta. Si parlava di pace, di solidarietà, di partecipazione, di riduzione delle servitù militari; tutti impegni sistematicamente disattesi con continui camuffamenti, rinvii, espedienti linguistici, rimpalli di responsabilità: una condotta che non si addice esattamente ad un Governo autorevole al quale preme il rapporto con i propri cittadini. La vicenda della base di Vicenza riassume didascalicamente questa strategia della "cortina fumogena". Per lunghi mesi, il Governo, messo alle strette dalla grande mobilitazione popolare, ha evitato di decidere, assicurando tuttavia due cose: che avrebbe tenuto nella massima considerazione le istanze della comunità locale e che nessun accordo formale autorizzava gli USA a entrare al Dal Molin, ragion per cui era possibile riconsiderare la scelta fatta dal precedente Esecutivo. Lo stesso ministro Parisi mise per iscritto, in una lettera indirizzata a me e ad altri senatori al tempo del rifinanziamento della missione afghana, queste cose, nel contesto di un *gentlemen agreement* - pensavo, un rapporto tra gentiluomini, ma purtroppo non è stato così - che prevedeva anche un significativo ridimensionamento delle strutture militari presenti sul nostro territorio, in particolare in quella terra martoriata che è la Sardegna che a lui, almeno quanto a me, dovrebbe essere particolarmente cara. Oggi, purtroppo, constatiamo che quell'accordo è carta straccia. Con un improvviso guizzo muscolare, il Presidente del Consiglio ha emanato un nuovo editto di Sofia, che dà il via libera agli americani, sulla base di motivazioni caotiche e contraddittorie, alludendo prima a misteriosi patti da onorare e invocando i supremi interessi della difesa nazionale, per liquidare poi la decisione come la più innocua delle scelte urbanistiche. Il ministro Parisi, per la verità, ha successivamente ribadito che patti da onorare non ce ne erano, avventurandosi per strade decisamente surreali, aggettivo usato spesso in Aula oggi. ha detto: «Gli americani avranno la base perché hanno presentato un progetto» (sembra interessante come decisione), attribuendo quindi la responsabilità della scelta al Governo in carica. Ma tutto ciò a questo punto non conta. Siamo di fronte alla rottura unilaterale di un patto collettivo sottoscritto con i cittadini tutti e con la comunità vicentina e di uno soggettivo stipulato con alcuni parlamentari, tra i quali il sottoscritto. È un fatto grave e doloroso, che azzera il dibattito di questi mesi e impone delle considerazioni conclusive. La prima è che il Governo, autorizzando la base al Dal Molin, ha fatto una scelta di guerra: ha deciso di assecondare una strategia fallimentare, quella della guerra preventiva, che ha disseminato di morte il pianeta e lo ha reso enormemente più insicuro; una strategia all'interno della quale le basi militari svolgono un ruolo insostituibile perché da esse partono gli uomini e i mezzi diretti in Iraq, Afghanistan e, nelle intenzioni di Bush (così è scritto nell'ultimo rapporto USA), in Iran, Siria e Corno d'Africa. Ogni base presente sul nostro territorio è un avamposto di guerra e questo è il ruolo affidato anche a quella di Vicenza. La seconda è una scelta contro la sicurezza dei cittadini. Ogni base militare comporta l'insediamento di armi micidiali (come i 90 ordigni nucleari presenti nel nostro territorio), esercitazioni belliche, incidenti di ogni tipo. Convincete la gente di Ghedi e di Aviano che le bombe atomiche che hanno sotto casa servono a proteggerli da Bin Laden e andate a dire a quelli di Quirra e Capo Teulada che i poligoni sono lì per la loro sicurezza, che le migliaia di bombe che finiscono in mare durante i giochi di guerra servono a incentivare l'economia della Regione, che le enormi porzioni di territorio espropriate e desertificate servono a proteggere l'ambiente. Anche su quest'ultimo punto non posso non sottolineare le promesse tradite. Non solo le servitù militari non sono state ridotte, ma quelle esistenti vengono ampliate, come a Vicenza, Sigonella, Quirra. Lo stesso calendario delle esercitazioni, che il ministro Parisi aveva assicurato sarebbe stato ridimensionato in Sardegna, non subirà alcuna limitazione. È notizia di ieri che per che per "superiori esigenze di difesa dello Stato" continueranno i micidiali bombardamenti aerei sulle spiagge di Capo Teulada e Capo Frasca, con buona pace dei pescatori, con buona pace dei pescatori, che da anni chiedono una tregua delle esercitazioni che consenta loro di pescare. Questo insieme di considerazioni spero serva a far capire che la scelta di autorizzare una nuova base militare ha implicazioni molto più complesse di quelle che solitamente vengono richiamate per giustificarne l'insediamento (problemi di difesa, di alleanze, urbanistici). Esse investono, al contrario, la sovranità territoriale, la difesa dei beni comuni, le dinamiche della rappresentanza e della partecipazione, dal basso, alla gestione del territorio. Lungo questo delicatissimo crinale si sta consumando una frattura profonda con l'autonomia del politico.

il giudizio che formuliamo in merito all'informativa qui svolta dal Ministro della difesa non può che essere nettamente negativo. Ribadiamo in questa sede le motivazioni che ci hanno condotto, in tutte queste settimane, ad esprimere la nostra nettissima contrarietà al progetto di raddoppiare la base militare americana Ederle nel territorio di Vicenza. Vorrei, infatti, ricordare che di questo stiamo parlando. Lungi dall'essere una questione «urbanistica», come il Presidente del Consiglio l'ha definita nelle settimane scorse, cercando di ridimensionare l'enorme gravità del suo assenso al progetto, la costruzione della base militare Dal Molin di Vicenza è uno dei perni di una politica aggressiva che gli Stati Uniti tentano di produrre sull'intero scacchiere mondiale, installando loro avamposti nel nostro Paese. L'Italia - e la base di Vicenza - come retrovia in cui insediare mezzi e armamenti per intervenire su un'area del mondo in cui si trovano 91 Paesi, tra l'Europa e la zona del Caucaso, la zona del Caspio, il Medio Oriente e tutta l'Africa. La 173a Brigata diventerà la più importante unità aviotrasportata e la più grande forza di risposta rapida alle dipendenze del Comando Usa in questa parte del mondo. Questo in un momento in cui la *leadership* americana non fa mistero di puntare sulla guerra - su nuove guerre - per puntellare il proprio sistema internazionale di potenza, pianificando appunto nuove *escalation* belliche, come in Iran, e rafforzando le tragiche occupazioni militari in corso, come in Iraq e in Afghanistan. Il fatto politico, di enorme gravità, di fronte al quale siamo posti è che il nostro Governo (e sottolineo il nostro Governo, perché ha vinto le elezioni anche grazie alla mobilitazione elettorale di centinaia, di migliaia di donne e di uomini che hanno costituito in questi anni il movimento per la pace) ha accettato supinamente una decisione del Governo degli Stati Uniti, funzionale alla politica estera di guerra preventiva e permanente, che in questi anni ha alimentato il terrorismo e la tensione internazionale e che è apertamente contestata, ormai, anche dalla maggioranza dei parlamentari e delle popolazioni nordamericani. Vi è poi un elemento altrettanto significativo, che attiene alle modalità con cui è stata condotta questa vicenda da parte del Governo. In pieno contrasto con il programma dell' Unione, dove si parla di coinvolgimento delle popolazioni locali, si è deciso senza tener conto del parere della popolazione di Vicenza, in larghissima parte contraria, come ci dicono tutti i sondaggi, l'ampliamento della base. Lo metto in evidenza perché lo stesso presidente Prodi ha recentemente criticato il Governo Berlusconi per non avere coinvolto l'opinione pubblica nelle trattative con gli Stati Uniti d'America. Giusto, ma quale coinvolgimento ha messo in atto il nostro Governo? Se noi ascoltassimo realmente la volontà della popolazione vicentina, ci accorgeremmo immediatamente dell'errore commesso. Avremmo la dimostrazione più nitida di come si sia scelta una strada per nulla rappresentativa del volere della comunità locale. Non solo, quindi, per nulla rappresentativa della volontà politica di milioni di elettori che hanno votato l'Unione per voltare radicalmente pagina, anche sul piano della politica estera. Per nulla rappresentativa della più complessiva volontà popolare. È possibile rimediare a questo grave *vulnus,* a questa lacerazione tra le ragioni del nostro popolo e le scelte del nostro Governo? Noi riteniamo che sia possibile a patto che si rimetta al centro del percorso di decisione, attraverso la consultazione referendaria vincolante, la cittadinanza di Vicenza e le forze sociali, politiche, le associazioni, le reti della società civile che in questi mesi si sono espresse, con straordinaria univocità, contro la costruzione della base Dal Molin. Noi sosterremo questa lotta, a partire dalla manifestazione del 17 febbraio, fino a quando la decisione non verrà rivista. Noi rimarremo fino alla fine al fianco del movimento contro l'ampliamento della base più. Il Governo deve saperlo. Concludo, signor Presidente, affermando che riteniamo sia giunto anche il momento di far conoscere al Parlamento e al Paese gli accordi segreti siglati con gli Stati Uniti negli anni '50 a proposito della presenza di basi americane nel nostro Paese. Occorre regolarizzare l'intera materia sulla base dell'articolo 80 della Costituzione, che impone la ratifica parlamentare sui trattati che comportano una cessione di sovranità. Affermo ciò poiché in questo contesto si inserisce, sicuramente, anche la base di Vicenza. Per queste ragioni, chiediamo ancora una volta al Governo di rispettare il programma dell'Unione, che non contempla affatto questo provvedimento, e la volontà della popolazione vicentina. E per queste stesse ragioni annunciamo sin d'ora che qualsiasi sia il proseguimento di questa vicenda noi continueremo la nostra lotta, a fianco del movimento per la pace per impedire l'ampliamento della base. *(AN)*. Signor Presidente, prima di entrare nel merito del discorso dell'allargamento della base per la 173a Brigata paracadutisti a Vicenza, mi piace cogliere un aspetto politico che paradossalmente si è verificato questa mattina: da questa parte vi è l'opposizione, che chiaramente denuncia certe carenze del Governo ed esorta il Governo a comportamenti coerenti in campo nazionale ed internazionale; dall'altra parte, sul Governo sono piovute una serie infinita di critiche, al punto che ci si chiede quale sia la maggioranza che regge questo Governo, cioè dove sia la maggioranza di Governo.

così come scompare una grossa parte dei rappresentanti della maggioranza e sul povero ministro Parisi e sui poveri Vice ministro e Sottosegretario piovono una serie infinita di critiche che mi fanno rivivere nei cinque anni scorsi. Ha ragione il senatore Colombo: che cosa stiamo facendo qui? Stiamo parlando di un Governo che ha un sostegno

responsabilità per carità di patria, ma è anche vero che credo sia giunto il momento che anche noi riflettiamo un po', perché non possiamo continuare a consentire che costoro governino un Paese e facciano una politica estera che è quella che si deve fare - sostenuti da noi. Ma quando mai? In quale Paese accade questo? Quello di stamattina è addirittura un fatto clamoroso e paradossale. Entrando nel merito del discorso,

«l'Espresso», con un articolo che raccontava un sacco di fandonie e di bugie, assolutamente non vere, ma che inquinarono la coscienza e la conoscenza dei cittadini di Vicenza. Fece eco a questo l'atteggiamento, che oggi abbiamo visto confermato, dei partiti dell'estrema sinistra e anche di una parte dei DS, naturalmente ancora una volta raccontando bugie, inesattezze, inesatte,

«È stata fatta la scelta della guerra». Ma per carità di Dio, lasciate perdere queste ridicole affermazioni, sulle quali avete lucrato per cinque anni, imbrogliando i cittadini italiani.

Questa è la democrazia che costoro intendono! Questo il modo di essere democratici che costoro intendono! Dall'altra parte c'è il Governo, il quale ha tentennato, ha traccheggiato, ha chiesto al Comune una cosa che non lo riguardava direttamente, non ha dato ascolto al Comitato paritetico; ha avuto paura delle manifestazioni che i suoi avversari interni continuavano a portare avanti, fino a quando ad un certo punto - siccome in politica estera non si possono raccontare le balle che si raccontano in politica interna pressato dagli americani che, gli hanno detto: «Amico mio, o ci dici di sì o ci trasferiamo completamente da Vicenza». Quello sarebbe il grave danno per la città di Vicenza, non la presenza degli americani: 750 posti di lavoro perduti, di un miliardo di euro per i lavori, di più di 200 milioni di indotto ogni anno. Quelli sarebbero i gravi danni che deriverebbero dall'andata via degli americani. L'unico danno dell'allargamento della base è rappresentato dalle manifestazioni che vengono sistematicamente condotte da questi forsennati che procurano solo disturbo alla città di Vicenza, la cui popolazione è - secondo recenti sondaggi, fatti da giornali seri che voi apprezzate, come il «Corriere della Sera» ed altri per cento favorevole all'allargamento della base. Allora, di che cosa venite cianciando sulla questione di sentire l'opinione? Siamo in democrazia; più del 60 per cento si dichiara favorevole, il Governo si dichiara favorevole, di quel Governo fate parte e, allora, fatemi la cortesia di finirla con queste manifestazioni gratuite che portano solo disturbo ai cittadini di Vicenza; parlo anche come senatore del Veneto, di uno che conosce le cose, caro amico onorevole Colombo. Attenzione, noi conosciamo la situazione; quando lei mi viene a raccontare di colate di cemento, la informo che nello stesso periodo in cui è prevista la realizzazione della base americana, in precedenza, a Vicenza sono state fatte dieci volte le colate di cemento per realizzare nuove abitazioni senza che nessuno abbia detto nulla. Quando mi si parla di un intervento che squilibrerebbe l'interno di Vicenza, occorre considerare che verranno 1.600 persone in

Abbiamo allora presentato questa mozione per chiedere al Governo - che è stato tentennante, che ha tirato fuori frasi come «non ero a conoscenza» o «non ne sapevo niente», che a un certo punto è risultato completamente spaccato nella sua maggioranza - una parola chiara, che in parte è stata già detta dal Ministro della difesa, al popolo italiano, una parola chiara agli alleati americani e anche una parola chiara e decisa a quella parte della sua cosiddetta maggioranza che continua a fargli la fronda. Il secondo aspetto, e concludo, è rappresentato, oltre che dal consiglio al Governo di tenere conto nelle trattative con gli americani della tutela dell'ambiente e delle ripercussioni sul sociale che potrebbero verificarsi

della nostra offerta, la facoltà di rivedere il regime dei dazi che penalizza l'industria orafa vicentina nei confronti di altri Paesi,

Da molto tempo a Vicenza si parla, tra vicentini e americani, dell'apertura di un istituto universitario politecnico, che sarebbe molto apprezzato da entrambe le parti. Ecco, dite agli americani di *speed up*, di accelerare la costruzione di questo istituto e allora la venuta della brigata non sarà, come qualcuno stupidamente ha detto, una scelta di guerra, ma sarà un ulteriore miglioramento della situazione della città di Vicenza.

il primo firmatario è la proiezione della necessità del nostro Paese di capire qual è il quadro politico italiano oggi, perché è sulla politica estera che si costruisce l'identità di un Paese, la sua credibilità internazionale. E su questo il Governo, purtroppo, non ha un itinerario chiaro, non ha un comportamento univoco,

determinate pubblicamente, fra i suoi esponenti autorevoli, fratture inemendabili. È l'eterno contrasto tra la sinistra antagonista e le altre componenti governative, che è la riprova che la coalizione elettorale non è riuscita a

che si sono lamentati del non rispetto da parte del Governo del loro programma. Ma non poteva che essere così, perché il Governo Prodi è figlio di un'alchimia politica, è figlio di alleanze improvvisate e così sull'allargamento della base di Vicenza il sì di Prodi, il sì di D'Alema e il sì di Parisi hanno trovato una ferma opposizione della sinistra radicale. Una parte del Governo si è dissociata pubblicamente, fino a definire uno schiaffo - come è stato detto ieri - il sì di Prodi a Vicenza. Gli impegni assunti a livello internazionale con Paesi alleati, per parte di questo Governo, nulla valgono rispetto al richiamo ad un pacifismo ad oltranza, rispetto ad un concetto di pace per la pace che sta costituendo un demagogico elemento di disinformazione dell'opinione pubblica, perché a Vicenza non si prevedono depositi di armi. *(Applausi dal Gruppo* *FI)*. E questi impegni assunti a livello internazionale nulla valgono anche rispetto alla volontà di segnare elementi di discontinuità nei confronti del Governo precedente, come se la guida dello Stato potesse avvenire e potesse andare avanti a segmenti. Noi chiediamo chiarezza, noi chiediamo che venga restituita al nostro Paese quella credibilità internazionale portata dal Governo Berlusconi. Siamo stanchi di assistere a dibattiti e a confronti fra le variegate componenti di questo Governo, che si riducono in realtà ad una costante opera di compromesso, relativa ad un'unica questione: come salvare il Governo cercando di rattoppare alla meglio tutte le falle che si aprono rispetto alla sua credibilità. Io credo che oggi Prodi debba prendere atto che la compagine governativa non può più considerarsi rappresentativa, né verso le istituzioni, né verso i cittadini, né del nostro Paese all'estero. Noi ci troviamo tra l'incudine di un Governo strenuamente attaccato al potere ed il martello di una politica ambigua e contraddittoria come quella di Vicenza, che rischia di far scivolare l'Italia verso le paludi di conseguenze catastrofiche sotto il profilo internazionale. Spesso, signor Presidente, si definisce questo periodo politico quello della Seconda Repubblica, ma io credo che, vista la situazione caotica in cui permanentemente versa, sia più esatto definirla come quello della Repubblica dei secondi!

nelle quali esprimiamo le nostre ragioni di contrarietà all'allargamento della base di Vicenza. Come ha ben sottolineato nel suo intervento il senatore Furio Colombo, chi si esprime contro l'ampliamento della base di Vicenza non mette in alcun modo in discussione - vorrei dirlo rispetto ai toni che ho sentito questa mattina negli interventi della destra - l'alleanza con gli Stati Uniti d'America. Non è questo il punto: il punto è come si sta nell'alleanza. Essa non ci obbligava e non ci obbliga affatto ad assentire alla decisione di trasferire a Vicenza la Brigata aeronavale, attualmente stanziata in Germania. Abbiamo sentito stamattina dall'esposizione un po' burocratica, per la verità, del ministro Parisi che la ragione della decisione presa in maniera affrettata è una richiesta dell'ambasciatore Spogli

sull'ipotesi di allargamento della presenza militare USA; la Commissione esteri del Congresso ha chiesto di fermare ogni rafforzamento della presenza militare USA nella zona, prima che si sia risolta la questione dell'Iraq, ma non vorrei che i colleghi della destra accusassero di antiamericanismo la maggioranza delle Commissioni esteri del Congresso degli Stati Uniti d'America. Credo che sia un modo vecchio di stare nell'alleanza quello di assentire rapidamente perché ci viene comunicato che vi è un certo passaggio parlamentare nel Congresso degli Stati Uniti d'America. Ci sono aspetti rilevanti che il Parlamento ha il dovere di discutere con serietà e senza strumentalizzazioni; vi è il problema del rapporto unilaterale

Il recente accordo Berlin Plus pone il tema di una sempre maggiore gestione europea delle basi dell'Alleanza. Non mi pare che la decisione presa dal Governo italiano vada in questa direzione.

Per questo mi ero permesso di chiedere un ulteriore chiarimento al ministro Parisi (è nello stampato). Quali sono gli accordi tra Italia e Stati Uniti che regolano lo statuto giuridico della base di Vicenza? Questi accordi sono tutti a conoscenza del Parlamento o ci sono clausole segrete? E soprattutto, nel momento in cui notizie quotidiane ci informano che vi è il rischio di un attacco militare verso l'Iran, con la dislocazione della flotta navale USA nel Golfo Persico, di ascoltare - che prevedono la codecisione del Governo italiano o almeno il suo consenso preventivo sull'uso delle basi

Chiediamo al Governo di sapere se non ritenga che debba essere rivisto lo statuto giuridico delle truppe americane operanti in Italia. Tutti ricorderanno la tragedia del Cermis; ci fu un'iniziativa meritoria del Governo italiano, ma il risultato fu quello della sottrazione del caso alla giurisdizione italiana. Infine, e mi affido alla sua sensibilità di uomo di sinistra, perdura lo scandalo della mancanza di libertà sindacale per i lavoratori italiani nelle basi USA, Sigonella e non solo. Da Ministro del lavoro posi il tema per la CGIL, ma anche per l'UGL, perché quella discriminazione, che risale ai tempi della guerra fredda, impedisce di fatto ai lavoratori italiani che operano in quelle basi di esercitare i propri diritti di libertà sindacale. Ci sono novità? È considerato irrilevante tutto ciò o o è più rilevante rispondere immediatamente alla richiesta di un ambasciatore, in vista di un voto nel Congresso degli Stati Uniti d'America che si terrà a giorni? Il secondo punto riguarda la visione burocratica della comunità locale ribadita nell'esposizione odierna del ministro Parisi. Faccio un richiamo al programma dell'Unione, il quale evidenzia in questo campo

Quindi, signori del Governo, è stato commesso un errore sul piano della democrazia, che deve essere alla base di ogni nostra iniziativa nel rapporto con le popolazioni locali. C'è una discontinuità negativa nella politica estera dell'attuale Governo,

in Africa, e questo sta già creando all'Italia problemi molto seri nelle sedi internazionali. In conclusione, credo che già dal 17 febbraio a Vicenza si farà sentire, come altre volte nella recente storia italiana, la voce del movimento per la pace, la voce che rappresenta la maggioranza degli italiani di ogni schieramento e certamente la larghissima maggioranza di coloro che ci hanno dato il consenso per governare. Questa voce e questo movimento potranno aiutare il Governo a ricondurre la sua azione su linee di fondo dalle quali queste recenti decisioni lo hanno purtroppo allontanato.

scontate, ma sono forse utili. Non c'è stato in questo dibattito un conflitto ideologico o di principio, non ci si è divisi sul sì e no alla NATO, sul sì e no

Non discutiamo, dunque, di un conflitto ideologico, ma possiamo discutere - e discuterne molto - sulle regole che riguardano gli impieghi operativi delle forze americane nella base di Vicenza, sull'utilizzo, in definitiva, della base. argomento il ministro Parisi ha detto qualche cosa di molto preciso che vorrei ricordare: «Sarà dovere del Governo assicurare la massima vigilanza circa il rispetto degli accordi bilaterali in materia di utilizzo della base per quel che riguarda gli impieghi operativi». operativi». Queste osservazioni vanno tenute nel giusto conto perché non sono casuali. Ad esempio, si potrebbe riflettere se sia - a me sembra non lo sia utile ed accettabile la presenza di armi atomiche nella base di Vicenza. Ad esempio, si potrebbe discutere di quello che l'ex ministro Salvi ha osservato circa i diritti sindacali ed altro ancora. Un'osservazione che penso si debba fare a proposito del dibattito che c'è stato è che non si devono mai confondere gli Stati con i Governi: si può essere critici su molte scelte del Governo Bush e, nel contempo, essere leali con l'alleanza rispetto agli Stati Uniti. Come si sa, i Governi passano, gli Stati restano e restano le linee di base della politica estera. Molti qui sono stati, sono e saranno critici verso il Governo Prodi e lo sono stati verso il Governo Berlusconi, ma tutti sono stati leali verso l'Italia. La lealtà verso la NATO non è in contraddizione con la critica verso alcune scelte dell'amministrazione Bush, anzi: più si è membri affidabili di un'alleanza, più si può, all'interno dell'alleanza stessa, far valere le proprie posizioni e ragioni. In questo dibattito è aleggiato un problema di fondo che certo non risolveremo oggi e non risolveremo da soli. È un problema che spesso solleva proprio il senatore Andreotti, che è un padre fondatore della NATO:

Oggi abbiamo problemi drammatici, ma profondamente diversi e quindi, forse, è giunto il tempo di aggiornare, con una lunga riflessione, il Trattato. Bisogna ascoltare le ragioni locali - è giusto che sia così - e bisogna concertare, bisogna ascoltare le critiche, che sono sempre legittime e che spesso possono far riflettere, però, alla fine, sempre, è compito della politica quello di decidere. Chi rappresenta le Regioni, chi rappresenta gli argomenti delle comunità locali? Io penso che le rappresentino la Regione, il Comune e la Provincia, che si sono pronunciate nella forma e anche nella sostanza. Ci si potrebbe semmai stupire perché, per una volta, in questa circostanza non è valsa la logica NIMN; *not in my neighbours*, non nei dintorni di casa mia. Le istituzioni si sono pronunciate secondo una logica diversa. Bisogna guardare la vicenda della base di Vicenza anche nel suo contesto generale. Noi non ci troviamo all'interno di una politica rivolta all'accrescimento della militarizzazione del territorio nazionale; al contrario,

alla Maddalena non ci saranno più militari americani e l'apparecchiatura sarà completamente smantellata. Sappiamo che la base della Maddalena pesa molto, ma molto di più di quanto pesi l'ampliamento della base di Vicenza. che la maggioranza è costituita da una coalizione di partiti. Se fosse composta da un solo partito, come in Gran Bretagna, ci sarebbero ugualmente, probabilmente, dei contrasti all'interno su temi come questo. Se la maggioranza fosse di centro-destra, ugualmente ci sarebbero dei contrasti - e ci sono - sul tema di Vicenza. Non ci si può dunque stupire del fatto che ci siano opinioni diverse di fronte a una scelta che ha un grande impatto ambientale e psicologico. Le obiezioni e le posizioni diverse vanno ascoltate tutte con rispetto, senza un processo alle intenzioni, senza cioè tacciare come antiamericane o pregiudiziali le posizioni di riserva e ostilità nei confronti dell'ampliamento della base. Concludo con un'ultima considerazione sul dibattito che si L'opposizione è costituita da grandi tattici e anche - mi si consenta - da grandi umoristi. Abbiamo ascoltato critiche dure nei confronti del Governo e le abbiamo ascoltate con rispetto.

Presenta un ordine del giorno che approva l'operato del Governo. Anche per queste ragioni, penso che il Governo possa imitare volentieri su questo terreno l'opposizione,

l'ordine del giorno presentato dalla maggioranza di Governo, il quale, tra l'altro, riproduce alla lettera ciò che è contenuto nel programma del Governo stesso.

Calderoli e Alberti Casellati e voteranno contro l'ordine del giorno presentato dalla maggioranza. Non possiamo non sottolineare il carattere paradossale di quanto sta avvenendo oggi con queste votazioni

mentre l'ordine del giorno di maggioranza prende solo atto delle dichiarazioni del Governo e lo impegna su una serie di temi che non hanno nulla a che vedere con il merito della questione che stiamo discutendo e con la decisione che il ministro Parisi ci ha illustrato questa mattina. Questo perché vi è un conflitto esistente all'interno della maggioranza, che è stato confermato dal dibattito. Non a caso il senatore Colombo ha parlato di solitudine del ministro Parisi rispetto alla sua maggioranza e il senatore Salvi ha definito la sua esposizione come un'esposizione meramente burocratica. Vi è un conflitto, ed è un conflitto che ha caratterizzato tutto l'atteggiamento del Governo in questa vicenda; un atteggiamento contraddittorio, contraddittorio, evidenziato proprio dalla ricostruzione precisa dei fatti che è stata svolta questa mattina dal ministro Parisi.

il pronunciarsi a favore o contro l'allargamento della base di Vicenza e che non era stato precostituito dalla maggioranza precedente alcun parere favorevole del Comune di Vicenza o del comitato paritetico della Regione, perché questi pareri sono arrivati, rispettivamente, nel giugno 2006 nell'ottobre 2006, cioè quando era già in carica l'attuale Governo. È chiaro che il tentativo di di trincerarsi dietro alle scelte degli enti locali - con quell'improvvida dichiarazione del presidente Prodi che ha detto: «Chi sono io, il sindaco di Vicenza?», come se questa fosse materia di competenza comunale comunale - maschera una contraddizione sulle decisioni che riguardano la continuità della nostra politica estera, dei nostri rapporti con gli Stati Uniti non l'eredità del precedente Governo, né possono essere evase rifugiandosi nelle competenze locali. È di tutta evidenza come il ricercare una via di fuga dalle responsabilità che spettavano al Governo è una strada che non poteva essere percorsa e alla fine il Governo ha dovuto assumersi le sue responsabilità, evidenziando il conflitto che divide questa maggioranza, che non è tra chi ha maggiore o minore sensibilità rispetto alle attese delle popolazioni locali, ma tra chi vuole mantenere una linea di fedeltà alla politica tradizionale di solidarietà euroatlantica e al sistema di alleanze del nostro Paese e chi invece risente di un antiamericanismo ideologico. Non si infatti, solo di un giudizio negativo sulla politica del presidente Bush, ma di un antiamericanismo ideologico, che ritiene di esprimersi con il «no» all' ampliamento della base militare di Vicenza per poi mascherarsi la dichiarazione di voler interpretare il sentimento delle popolazioni locali. In realtà, dietro questa dichiarazione c'è solo il tentativo di coprire le contraddizioni di questa maggioranza su un tema cruciale per il nostro Paese, quale quello della politica estera. Una maggioranza incapace di una coerente linea di politica estera è una maggioranza che il nostro Paese non merita.

della maggioranza, che scaturisce dopo una serie di difficoltà oggettive su una materia che va ad incidere direttamente su una fascia importante di popolazione che ha manifestato e manifesta, per certi aspetti, contrarietà a questa decisione. Non sarei onesto con me stesso e con il Gruppo che rappresento se non dicessi che arriviamo a sottoscrivere questo atto con molta difficoltà,

Difficoltà però che, con spirito di solidarietà, abbiamo superato all'interno del nostro ragionamento, per non far mancare il nostro contributo nella direzione del miglior esito complessivo possibile di questa vicenda. I senatori dell'Italia dei Valori, voteranno

Signor Presidente, onorevoli colleghi, a nome del Gruppo Per le Autonomie, dichiaro fin d'ora che voteremo contro tutte e tre le mozioni presentate dall'opposizione. Sono strumentali e non hanno altro scopo che scomporre la maggioranza, creare nuove alleanze e quindi far cadere il Governo. Voteremo invece con convinzione l'ordine del giorno presentato dai Capigruppo di maggioranza, che tiene conto e rappresenta una sintesi delle sensibilità e delle preoccupazioni del Paese che hanno trovato voce in tante dichiarazioni svoltesi in quest'Aula da parte degli esponenti dell'Unione. Esso rispecchia *in toto* il programma dell'Unione prevedendo una conferenza nazionale sulle servitù militari alla luce anche dei timori espressi dalla popolazione locale. Ritengo comunque che la vicenda della base di Vicenza debba offrire lo spunto per accelerare nel nostro Paese, come negli altri Paesi europei, un processo di riflessione profonda e di ripensamento su ruolo e compiti della Nato. L'Alleanza Atlantica - come è noto - è nata nel 1949, all'inizio della cosiddetta Guerra fredda. Nella logica dei due blocchi contrapposti, la NATO doveva difendere l'Occidente dal presunto attacco da parte dell'Unione Sovietica e dei Paesi dell'Est che facevano parte del Patto di Varsavia. La caduta del muro di Berlino, il crollo dell'Unione Sovietica e il dissolvimento dei regimi comunisti negli Stati dell'ex «cortina di ferro» ha di fatto mutato radicalmente gli scenari internazionali e conseguentemente le politiche da seguire. Dopo l'11 settembre è la lotta al terrorismo la sfida principale da affrontare. Si tratta di una sfida globale alla luce della quale ritengo che anche i ruoli delle alleanze internazionali debbano essere ripensati. Nel non disconoscere le responsabilità che al nostro Paese derivano dalla sua collocazione internazionale e dalle sue alleanze storiche, auspico tuttavia che il Governo avvii un ragionamento con gli Stati Uniti e all'interno della NATO sulle basi militari presenti sul nostro territorio e soprattutto sul loro utilizzo. L'obiettivo deve essere una nuova politica della pace, che cerca il consenso e non lo scontro delle civiltà, non le aggressioni belliche che purtroppo sono state portate avanti anche dalle nostre basi militari in Italia dal Governo di Bush (e non dico dell'America); devo essere il devo essere il dialogo e il confronto sui temi, cercando una soluzione di pace. Onorevole signor Presidente, sappiamo che nella base di Vicenza il generale americano è il comandante generale della SETAF (la *Southern European Task Force*) nonché comandante di tutte le forze americane presenti a Vicenza. Nell'ambito della SETAF opera una brigata paracadutisti USA che tre anni fa era impiegata in Iraq e successivamente in Afghanistan. Non possiamo accettare che, con l'ampliamento della base la caserma Ederle di Vicenza che, ospita appunto il comando della *US* *Army* per l'Europa del Sud, si corra il rischio che questa diventi il cervello di operazioni unilaterali statunitensi in Medio Oriente. Detto questo, ritengo che il Governo abbia gestito male la questione. Lo scorso 16 gennaio l'Esecutivo ha annunciato il suo sì all'ampliamento della base USA di Vicenza, affermando che la vicenda non rappresenta un problema di natura politica bensì una questione di carattere urbanistico-territoriale e che, pertanto, avrebbe seguito il parere del consiglio comunale di Vicenza che si era espresso a favore dell'ampliamento. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a mio avviso si è stati troppo superficiali e soprattutto poco trasparenti con la comunità interessata su un tema così delicato. Il Governo - sia l'attuale sia soprattutto, quello precedente - avrebbe dovuto coinvolgere maggiormente nella fase decisionale la popolazione interessata, perché è anche compito dell'Esecutivo centrale confrontarsi con le popolazioni locali quando si tratta di fare scelte che hanno un impatto così rilevante su un'area. Questa richiesta è stata fortemente proposta

In queste settimane le comunità della zona hanno fortemente manifestato la propria preoccupazione in ordine all'inquinamento acustico e ambientale, alla sicurezza, alla mobilità, alle infrastrutture e ai servizi e, anziché coinvolgerle attivamente nella fase antecedente all'annuncio della decisione presa dal Governo, abbiamo assistito soprattutto a tentativi di autoassoluzione tra il Governo centrale e quello locale. Sarebbe stato giusto - a mio avviso - accogliere la richiesta della popolazione di indire un *referendum* consultivo per assumere una decisione più condivisa. Ci auguriamo comunque che il Governo adempia al suo dovere di assicurare la massima vigilanza sul rispetto degli accordi bilaterali in materia di utilizzo della base stessa per quel che riguarda gli impieghi operativi; e che tenga costantemente e dettagliatamente informato il Parlamento sull'utilizzo dell'opera: non vorremmo che

La questione dell'ampliamento della base di Vicenza non può e non deve essere comunque connessa alla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali multilaterali e, nello specifico, al rifinanziamento della missione italiana in Afghanistan. Su questo delicato argomento, che avremo il compito di esaminare a breve, mi permetto soltanto di sottolineare, signor Presidente, l'urgente necessità di arrivare ad una conferenza internazionale di pace sull'Afghanistan nell'ambito delle Nazioni Unite, che raccolga intorno a un tavolo tutte le forze interessate di quell'area geografica per creare pace e non guerra. *(Applausi dai

nel febbraio del 1998 un aereo dei *marines*, di base ad Aviano, tranciò di netto uno dei cavi della funivia del Cermis. La cabina, con 20 persone, precipitò nel vuoto: nessun superstite. La corte marziale americana assolse il *marine* dall'accusa di omicidio e fu condannato a sei mesi di carcere. L'ho ricordato perché, durante quel volo, fu violata ogni regola sulla rotta, sulla velocità e sulla quota da tenersi. Non era il primo volo di quel tipo, badate bene, ma una prassi, una bravata che si faceva sempre e si ripeteva in occasione del trasferimento dei militari: una sorta di allegra onnipotenza per cui i *marines* si comportavano come se il nostro territorio fosse loro, considerandosi sopra le regole, onorevoli colleghi, veri e propri occupanti, tanto che i lavoratori italiani delle basi devono sottostare alle leggi americane. Una per tutte: vige ancora a Vicenza il più fiero maccartismo, tanto che i lavoratori non possono iscriversi alla CGIL, perché sono in odore di comunismo e, come voi sapete, il maccartismo non si è mai appannato nelle loro coscienze. La vicenda del Cermis, (ma non dimentico l'uccisione di Nicola Calipari per mano americana), mai seriamente indagata, mai chiarita, è una delle ragioni per cui siamo nettamente contrari al raddoppio della base USA. E voterò, con tutto il Gruppo, contro ogni mozione che ne prefiguri il raddoppio. L'Italia è diventata una portaerei statunitense: ci sono basi a Napoli, Sigonella, Gaeta, Maddalena, Aviano, Camp Darby e, appunto, a Vicenza. Sono già state ingrandite le basi di Aviano e Napoli-Capodichino e un'importante struttura per l'alloggio dei militari e dei familiari è stata realizzata a Gricignano di Aversa, così come sta avvenendo a Sigonella. Il Governo, il nostro Governo, farebbe bene a rivedere tutta la politica delle servitù militari, perché esse sono davvero un attentato alla sovranità del nostro Paese. E poi, che senso ha, dopo la fine della Guerra fredda? L'Italia non è più quel Paese di frontiera di grande importanza geopolitica. Perché permettiamo ad un Paese straniero di utilizzare quegli stessi spazi - ampliati, ristrutturati, ammodernati - in nome della cosiddetta guerra umanitaria? Una guerra che ha incattivito il mondo, signori del Governo, voi lo sapete, l'ha insanguinato, ha reso il terrorismo più forte, ha provocato, soprattutto, una pericolosissima inimicizia dei popoli del Medio Oriente nei confronti di noi occidentali. Sta qui lo stretto legame tra l'ampliamento di Vicenza e una guerra sbagliata, fallimentare, come quella in Afghanistan.

Entro il 2010, l'aumento sarà di circa 1.800 militari statunitensi. Dai 2.750 attuali, Vicenza ne ospiterà 4.500, un vero e proprio esercito, tutti superaddestrati e superarmati. Da lì quegli uomini statunitensi partiranno per bombardare l'Iraq e l'Afghanistan, e si parla del loro utilizzo nel caso di un attacco all'Iran. Sto dicendo,

Cresceranno i rischi perché gli italiani verranno considerati, a tutti gli effetti, sostenitori della politica di guerra di Bush, ci sarà un aggravamento della sicurezza nazionale. Ma questo non pretende una riflessione più attenta, una cautela più rigorosa? Non pretende, soprattutto, un coinvolgimento pieno, finora assolutamente disatteso, del Parlamento italiano? Negli Stati Uniti c'è una contestazione aperta alle guerre di Bush e al raddoppio delle basi, lo diceva il senatore Salvi ed ha ragione. E noi, che ce ne siamo andati via giustamente dall'Iraq, che ci siamo impegnati positivamente in Libano, raddoppiamo Vicenza, la militarizziamo, ne facciamo un'enorme portaerei militarestatunitense. Vorrei Vorrei una risposta, signori del Governo, che non ripetesse il rosario degli impegni internazionali che vanno rispettati, che non dicesse - come è stato detto - «nessuno se ne va, non possiamo andarcene noi» perché non significa nulla. E perché mai un Paese libero, autonomo, responsabile, non dovrebbe rifiutarsi di offrire agli Stati Uniti d'America un appoggio logistico a guerre sbagliate e nei fatti già perse? L'Iraq è un mattatoio. In Afghanistan i talibani e i signori della guerra sono più forti di prima, coinvolti nel Governo fantoccio di Garzai in prima persona e padroni dell'oppio. Guerre perse. Si può continuare a stare lì

Sulla questione israelo-palestinese, ad esempio, sul Libano, sulle critiche al carcere di Guantanamo. Non erano scontate, erano importanti. La scelta di Vicenza, però, rischia di rendere tutto questo vano. Chiedo al Governo di tener conto dell'ostilità dei vicentini, delle grandi preoccupazioni - per usare un termine non adeguato - della sua maggioranza, di rivedere la sua decisione per la sicurezza dei cittadini italiani e per il mandato di pace ricevuto dagli elettori. Sarebbe un atto di autonomia della politica dagli USA, contro l'appiattimento ad essa che ha caratterizzato il precedente Governo. E considero non accettabile il raddoppio della base USA di Vicenza senza che i problemi connessi - dalla sicurezza dei vicentini e degli italiani

signor Presidente, signori del Governo, è una democrazia parlamentare. *(Applausi

che andrò a descrivere non ne avevo mai viste e pensavo di non vederne. Chiederò al mio amico Peterlini in base a quale logica ha affermato che voterà contro un ordine del giorno che dice testualmente: «Il Senato, udite le comunicazioni del Governo, le approva». Questo è un ordine del giorno sul quale lo stesso Governo si è dichiarato contrario. Non riesco davvero a capire la logica. Qualcuno deve spiegarmela.

La 173a Brigata è già attualmente in parte di stanza a Vicenza e il suo comando è già a Vicenza.

i criteri di accorpamento sono stati studiati e presentati in uno stretto contatto coordinato dalle competenti autorità italiane, secondo le procedure usuali. Le nuove strutture, le attività dei militari, l'equipaggiamento previsti all'aeroporto

non vede più nessun militare italiano dell'Aeronautica di stanza: ci sono solo dieci furieri per la manutenzione degli impianti,

La gestione della pista e di ogni struttura esistente nell'aeroporto resta di totale controllo e gestione delle competenti autorità militari italiane. Aviano, che già esiste, resterà il riferimento per ogni volo operativo della SETAF; i progetti di infrastrutture proposti all'esame e alle valutazioni della competenti autorità italiane sono stati studiati nel pieno rispetto e considerazione sia del tessuto urbano che dell'ambiente circostante, logicamente per limitare l'impatto ecologico, eccetera.

della cittadinanza vicentina, che va affrontato con il massimo rispetto. Chiedo quindi di creare un tavolo di concertazione per scambiare le nostre opinioni fra Governo, enti locali

Leggo testualmente: «Nelle ultime settimane si è assistito ad un singolare rimpallo di responsabilità su chi debba prendere una decisione relativamente alla realizzazione delle nuove infrastrutture, con l'amministrazione comunale vicentina». Ma, l'amministrazione comunale vicentina ha solo un potere consultivo: è questo Governo che deve decidere e doveva decidere prima!

è stato veramente utile portare il dibattito sulla base di Vicenza nella sua sede propria: in Parlamento e al Senato. Devo dire che il dibattito è stato interessante e ha portato molti elementi di novità e di chiarificazione. Abbiamo sentito il senatore Salvi parlare come il *leader* di un partito nuovo:

registrato un Governo - mi scusi il vice ministro Intini, a cui va tutta la mia umana simpatia - costretto a negare l'evidenza; cosa che, forse per motivi di carattere sardo, il ministro Parisi si è rifiutato di fare e, infatti, non c'è. Come si fa infatti a dire che tutta la maggioranza è d'accordo sulle linee fondamentali della politica estera del Governo? La base di Vicenza è un caso di non grande importanza, ma che acquista un'importanza politica straordinaria in quanto è l'occasione perché si rivelino i segreti pensieri dei cuori; abbiamo ascoltato i segreti pensieri dei cuori della sinistra. C'è in Italia una sinistra comunista che è ancora convinta che Pol Pot avesse ragione e gli americani avessero torto, che Stalin avesse ragione e gli americani avessero torto, che è ancora convinta che gli americani hanno sbagliato a non permettere che in Italia ci fosse la rivoluzione comunista dopo il 1945 e alla fine della Seconda guerra mondiale. È questa infatti la colpa che voi rimproverate agli americani; la prima e fondamentale colpa che rimproverate loro. Abbiamo sentito accenti che era tempo che non ascoltavamo. Se fosse vera la metà di ciò che ha detto la senatrice Palermi, non solo non dovremmo permettere il raddoppio della base di Vicenza, ma dovremmo pretendere che gli americani chiudano la base di Vicenza immediatamente. Infatti, l'immagine che voi date è quella che al mondo la minaccia per la pace non viene dal terrorismo islamico, che non c'è una guerra contro il terrorismo: c'è un imperialismo americano che minaccia la pace dei popoli e l'Italia quantomeno deve rimanere neutrale per vigliaccheria, ma se avesse coraggio dovrebbe schierarsi col fronte imperialista contro gli americani. *(Applausi dal Gruppo* *UDC).* Come fa, signor vice Ministro, a dire che la sua maggioranza sostiene la sua posizione di politica estera sulla base di Vicenza o su qualunque altra questione? Ciò significa andare contro l'evidenza. Veniamo alle mozioni che sono sottoposte alla nostra attenzione. Qui il paradosso va veramente oltre il limite del ridicolo. L'opposizione è convinta che in politica estera i Paesi devono avere linee di lungo periodo, che la politica estera non può cambiare ad ogni elezione. Tra l'altro, è per questo che non ve la cavate dicendo che siete con l'America e contro Bush, perché le linee fondamentali di una politica estera vanno oltre i singoli Governi che di volta in volta la interpretano. sono fatte per durare decine di anni e il problema non è se oggi governa Bush in America e domani, chissà, Hillary Clinton o un altro: il problema è se l'America è una grande Nazione insieme alla quale condividiamo interessi, ma anche valori fondamentali e se siamo nella lotta contro il terrorismo insieme con gli Stati Uniti oppure contro gli Stati Uniti; se predomina per noi l'idea dell'imperialismo americano da combattere o di un terrorismo che è la grande minaccia per la pace e per i valori democratici. Tra l'altro, il fatto che la base di Vicenza sia una base retta da un accordo bilaterale Italia-Stati Uniti ci porta anche a chiedere un'altra cosa: cosa: quando parliamo di Unione Europea, la vogliamo dentro una comunità atlantica, dentro una più ampia solidarietà atlantica o la pensiamo in contrasto, in opposizione al resto della comunità atlantica, cioè agli Stati Uniti ed al Canada? Sono questioni fondamentali di politica estera alle quali non si sfugge. non ho ascoltato, signor Vice ministro, parole di simpatia, di comprensione o di sostegno per il suo Governo che non siano venute dall'opposizione.

ci va bene. E ciò non è paradossale, signor Vice ministro, ma corrisponde alla logica di un grande Parlamento democratico. È normale che l'opposizione, sulle grandi questioni di politica estera, aggiunga i suoi voti alla maggioranza. È una garanzia che si dà ai *partner* del Governo italiano che, quando cambierà il Governo

Ciò che non è normale è che la maggioranza non sostenga il Governo. E questo oggi, in quest'Aula, è risultato con limpida e cristallina chiarezza. Peterlini, non è il nostro ordine del giorno che tenta di dissolvere la coesione della maggioranza, siete voi che avete mostrato che la maggioranza non ha alcuna coesione sulla politica estera! E un Governo che non ha coesione in politica estera, non ha coesione, perché non si può governare un Paese se non si ha una visione della sua collocazione internazionale. Come dicevo, l'opposizione offre i suoi voti per permettere all'Italia di fare una degna politica estera, per mostrare che l'Italia è un *partner* affidabile,

atto vuol dire che forse una metà della maggioranza approverebbe le dichiarazioni del Governo, se avesse il coraggio di votare con l'opposizione (ma evidentemente non lo ha), e l'altra metà non le approverebbe; così ognuno rimane sulle sue posizioni. Per coprire questa assoluta inconsistenza politica, questa mancanza di unità,

il Governo «a dare impulso alla seconda conferenza sulle servitù militari, coinvolgendo l'Amministrazione centrale della difesa, le Forze armate, le Regioni e gli enti locali» - perché non anche le società bocciofile? - «al fine di arrivare ad una soluzione condivisa».

per dire che il Gruppo dell'UDC rivolge un appello al Presidente della Repubblica affinché svolga una funzione di alta suasione morale per convincere il Governo a presentarsi nelle Aule del Senato e affrontare un dibattito sulla politica estera che si concluda con una mozione che ci spieghi finalmente qual è la politica estera di questo Governo e di questa maggioranza. dal risultato di questo dibattito noi comprendiamo che il Governo ha una politica estera e la maggioranza ne ha un'altra, incompatibile ed incomponibile con quella del Governo.

voterà a favore dell'ordine del giorno della maggioranza unita; un importante ordine del giorno di respiro strategico, checchè ne dica il presidente Buttiglione, e contro la mozione chiaramente strumentale delle destre. ultima, infatti, ci parla di una politica internazionale ormai sconfitta, sconfitta nella dottrina della guerra preventiva globale, come nella crisi politica e di consenso del Governo Bush e del paradigma neocon. Lo faremo in nome della nuova politica estera italiana, che molto abbiamo condiviso e che Governo e maggioranza hanno ricollocato sull'asse della ricostruzione della autorevolezza delle Nazioni Unite, della soggettività politica europea, del multilateralismo dinamico, della strategia euromediterranea, sul piano della cooperazione e delle sinergie produttive. È per questo che riteniamo il raddoppio del Dal Molin un errore grave che pone in un cono d'ombra la stessa politica estera del Governo e contraddice il programma dell'Unione. Vi è qui, innanzitutto, una umiliazione democratica che offende, come hanno spiegato i senatori Valpiana, Brisca Menapace, Del Roio, Del Roio, Grassi. Siamo alla sconnessione tra rappresentanza e partecipazione, di fronte ad uno Stato che esalta la propria ragione separata da diritti e volontà delle comunità, rendendole mute ed invisibili. Sono negati sentimenti, affettività, intelligenze, saperi collettivi, rinchiusi in aree destinate ad essere recintate ed inviolabili come Guantanamo, come ha scritto non un bolscevico, ma Gian Antonio Stella sul «Corriere della Sera» e coperte da 700.000 cubi di cemento in una città preziosa; tutte cose che si sarebbero potute vedere, che nulla hanno a che fare con l'antiamericanismo. Bastava andare a Vicenza, ma nessuno è andato. Avrebbero visto, come ha scritto Ilvo Diamanti, nemmeno lui bolscevico, le famiglie borghesi vicentine, le donne, splendide protagoniste di quella resistenza, che difendono le proprie vite e le proprie abitazioni. Ma così, colleghe e colleghi, il potere diventa sfera separata, *élite* di regista, metafora autoritaria. È da qui che rischia di nascere la tanto temuta fuga dalla democrazia, l'antipolitica: la resistenza di massa, radicale, forte, non violenta delle comunità vicentine è per questo un atto di democrazia e un atto di alta politica. Noi ci sentiamo parte di questa resistenza; parte di queste comunità che si autodefinisccono, conflittualmente, nella cittadinanza di territorio. Siamo all'interno dei loro obiettivi e dei loro percorsi. Lotteremo insieme fino al mutamento della decisione del raddoppio; se sarà necessario, nel corpo a corpo

Affrontiamo un tema, infatti, non urbanistico ma squisitamente politico. La nuova base sarà il trampolino di lancio delle operazioni militari statunitensi inserite nella dottrina sconfitta della guerra preventiva globale. Per il nostro

generale è anch'esso a Vicenza, è stato trasformato da comando di appoggio logistico in comando di teatro, responsabile del ricevimento, della preparazione al combattimento e del movimento avanzato delle forze che entrano nella regione meridionale per una guerra». Questo è un documento del Dipartimento di Stato: la base allargata di Vicenza, collegata alle basi aeree di Aviano e di Sigonella e a quella logistica di Camp Darby, è un trampolino di lancio di operazioni militari. Ma vi è anche un altro tema, a questo punto, di alta politica istituzionale che vogliamo sottolineare: il Parlamento ed il Governo italiano non hanno alcun potere decisionale ora sulle operazioni militari statunitensi. Qui non c'entra la NATO, ma operazioni militari statunitensi, che, partendo dal nostro territorio, coinvolgono automaticamente il nostro Paese in guerre, neppure dal Parlamento e dal Governo decise. Siamo infatti ancora all'Accordo generale bilaterale stipulato il 20 ottobre 1954, il cui contenuto rimane riservato. Siamo ancora immersi nei segreti militari imposti dalla riservatezza dei patti militari durante la Guerra fredda. Non siamo nemmeno di fronte al Trattato NATO, ma a un trattato bilaterale mai portato in Parlamento per la ratifica. Ebbene, ci ricorda giustamente Spataro che i Parlamenti di altri Paesi che ospitano basi degli Stati Uniti (pensiamo alla Spagna, al Portogallo, alla Grecia, perfino alla Turchia) hanno discusso e deliberato sui trattati bilaterali. A quasi sessant'anni dal primo accordo bilaterale,anche è cambiato il mondo, è crollato il Muro di Berlino, si è sciolto il Patto di Varsavia, viviamo l'internazionalizzazione geopolitica della globalizzazione, l'Italia permane come nicchia di una nuova Guerra fredda, di un nuovo maccartismo dello Stato di eccezione democratica, imposto da un impero tanto più pericoloso perché in crisi. Chiederemo formalmente, in coerenza con il programma dell'Unione richiamato nell'ordine del giorno e come sviluppo della nuova politica estera del Governo italiano, la declassificazione dell'accordo del 1954 e di tutti gli accordi bilaterali ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione, che impone la ratifica parlamentare dei trattati che comportano una cessione di sovranità.

il popolo dell'Unione, il popolo che ha voluto e vuole questo Governo, perché corregga, ministro Parisi, vice ministro Intini, una decisione che è innanzi tutto incomprensibile, prima ancora che sbagliata.

Signor Presidente, la nostra mozione - rispondo al senatore Peterlini - mi sembra abbia avuto un grande significato, insieme alle mozioni di Forza Italia e della Lega: un dibattito che, devo dire, è stato estremamente interessante e le cui conclusioni (e mi stupisce il senatore Russo Spena, che spesso ho apprezzato per la coerenza e la moderazione con cui parla), dimostrano che evidentemente non si tratta di un atto di pubblica amministrazione, di un consiglio comunale o di una delibera di un assessore all'urbanistica. Abbiamo evidentemente toccato temi che hanno dilaniato e appassionato i partiti della coalizione di maggioranza. Forse la prima considerazione cui dobbiamo giungere è che il vero problema della nostra politica estera è che non è estera, cioè tratta di tutto fuorché di politica estera: è la solita cucina all'italiana di tanti sentimenti, di tante passioni, di tanti interessi *(Applausi del Gruppo AN)* e misura un ritardo culturale della sinistra antagonista,

che l'hanno portata a far parte della coalizione. Questo è l'errore di Russo Spena, che dimentica che non è qui a rappresentare solo e soltanto le formazioni pacifiste e i cittadini che intende rappresentare, ma che è un esponente della maggioranza e quindi

sostenendosi che in fondo questo era il vero problema, cioè come in qualche modo difendere gli interessi dei cittadini di Vicenza. Nel momento in cui, però, abbiamo presentato un ordine del giorno (su cui ritornerò) è riscattato il meccanismo che evidentemente avevamo provocato e, cioè, l'azione del Governo che, nella sostanza, gran parte della maggioranza non approva, tant'è che gli interventi della senatrice Palermi e del senatore Russo Spena di tutto hanno trattato fuorché di Vicenza (abbiamo sentito parlare del Cermis, dell'internazionalizzazione della politica estera, abbiamo visto partire la 173ª brigata per l'Iran prima ancora che abbiano dichiarato guerra). Il problema si è rispostato e il tentativo di ritornare a Vicenza è miseramente fallito in quest'Aula, dimostrando, ancora di più in questa sede, le differenze all'interno della coalizione. Caro vice ministro Intini, spesso ho apprezzato la sua serenità, però qualche volta la serenità di fronte a queste vicende equivale al non vedere quello che succede. Nel corso del dibattito, mi è venuta in mente una cosa che ho sempre molto apprezzato: se andate a Gibellina, la città distrutta dal terremoto, un grande scultore, Burri, l'ha coperta con delle lenzuola di cemento per nascondere cosa c'è sotto. Credo che questa mattina Burri sia stato in quest'Aula e abbia messo, o tentato di mettere, molte lenzuola di cemento sulle rovine di una maggioranza che vuole apparire all'esterno ancora un fatto

una serie di risposte estremamente precise quando, richiamando la questione delle procedure, ha anche ribadito che la posizione ufficiale del Governo era quella dell'alleanza con gli Stati Uniti, che non vi erano problemi di discussione dell'Alleanza e che il nostro sistema di alleanze era assolutamente garantito. Allora, è ovvio ed evidente che se veniamo in quest'Aula a porre una questione e il Governo risponde nella misura in cui noi abbiamo chiesto, non vi è nulla di ironico, nulla di scandaloso, nulla di provocatorio nel presentare un ordine del giorno che dice: si approvano le relazioni del Governo.

Gruppo AN).* Non abbiamo problemi. Ripeto: «il Senato della Repubblica, udite le comunicazioni del Governo, le approva in parte», perché questa è la sostanza. Non precisiamo la parte. Questa è la posizione. Vice ministro Intini, noi apriamo - credo - un caso nuovo nella storia della democrazia perché il rappresentante del Governo in quest'Aula respinge un ordine del giorno che approva l'operato del Governo.

In quale condizione vi siete messi nel momento in cui - ripeto - il Governo non approva l'ordine del giorno che approva l'operato del Governo?

del dibattito aperto tra le forze politiche e nell'opinione pubblica. Prende atto: siamo in una fase di dibattimento. Le dichiarazione di Parisi (che corrispondono a quella di Prodi, secondo cui la decisione su Vicenza il Governo l'ha presa ed è quella) vengono rimesse in discussione nell'ordine del giorno della maggioranza,

mi dicesse cosa è la conferenza nazionale sulle servitù militari, che è così importante da risolvere tutti i problemi della politica estera che abbiamo trattato in questa sede. Mi domando: nel momento cui verrà respinto l'ordine del giorno che approva l'operato del Governo e verrà approvato un ordine del giorno che prende atto dell'operato del Governo, il Presidente della Repubblica, di fronte a un tale atto, come si dovrà comportare? Cosa ne deve dedurre? Quale tipo di atteggiamento può assumere la più alta carica dello Stato quando il Senato della Repubblica vota contro l'approvazione della linea del Governo e quindi, sostanzialmente, sfiducia l'azione del Governo? Non è necessario, a questo punto, coprire questo *vulnus*, in qualche modo riaprendo un dibattito sulla politica estera, in modo che possa essere discussa serenamente e si possa uscire da questa cultura della cucina di casa, della maionese impazzita (per usare un espressione non mia, ma del presidente del Consiglio Prodi), e capire questa maggioranza che tipo di linea politica ha e che cosa approva del Governo? Di cosa prende atto?

del fatto che le basi americane possono essere usate senza consultare le comunità nazionali quando al Governo c'è D'Alema che decide di bombardare la Serbia e che quindi è proibito ai governanti di centro‑destra usare le basi americane senza l'approvazione della sinistra? dai Gruppi AN e FI)*. Di cosa prende atto questa maggioranza? Credo che vi siate infilati un terribile vicolo cieco, perché la figura peggiore in quest'Aula la fa la maggioranza, che non solo non approva la linea del Governo, ma dimostra di non essere coesa, di non essere in grado di reggere le responsabilità che derivano dalla politica estera di non essere capace di reggere le scelte e le decisioni di grande realismo e di grande responsabilità che impone la politica estera. Non si fanno le campagne elettorali e amministrative, non si fanno i congressi di partito con la politica estera! Questo lo fate voi. Noi, ci rifiutiamo di farlo.

Quante politiche estere? Forse più di una, anzi sicuramente più di una. Ma, poiché la politica è una scienza esatta, quando le coalizioni elettorali (e non politiche) sono chiamate a governare, tutti i nodi vengono al pettine, emergono le contraddizioni ed emerge la paralisi decisionale su quei temi dove vi era convergenza non politica, ma soltanto elettorale. Questo Governo raggiunge ormai la paralisi: è fermo sulla riforma delle pensioni, è fermo sulla riforma fiscale, è fermo su tanti altri temi, quali quelli etici, ed è paralizzato sulla politica estera. Lo scenario di oggi lo conferma: vota contro se stesso. Qui vi è in discussione, signor Presidente, un concetto forte: l'alleanza con gli Stati Uniti, vista come rapporto con l'Occidente nel contrasto al terrorismo e al fondamentalismo che attaccano e mettono in discussione la nostra libertà e la nostra democrazia.

Noi eravamo per la logica di un'attenzione al conflitto mediorientale che guardasse ad Israele come paese aggredito e non aggressore. Abbiamo un Ministro degli esteri che, invece, coniando l'espressione della "equivicinanza", sposta l'attenzione da Israele alla Palestina e all'Iran. Vorrei ricordare come, nel giro di sei mesi, abbia dimostrato fattualmente questa attenzione antisraeliana. In sei mesi il ministro D'Alema si è lasciato andare a dichiarazioni come: Gaza, reazione Israele non proporzionata; visione militare Israele accresce odio e insicurezza; con offensiva Israele si rischia; la posizione di Israele è insostenibile; grave errore Israele non cessare il fuoco; ed altro. Si guarda con attenzione, invece, a uomini emergenti dell'Iran, i quali la pensano in maniera diametralmente opposta, in chiave non soltanto antisraeliana, ma addirittura distruttiva nei confronti di quel Paese. Ahmadinejad dice che il destino di Israele è la distruzione; tolleranza tolleranza per tutti fuorché per Israele; Israele è destinato a scomparire; Israele scomparirà presto. Ebbene, dinanzi a queste dichiarazioni il nostro Ministro degli Esteri che cosa fa?

Si guarda quindi ad un baricentro ben diverso e differente rispetto a quello del passato. Nel Governo emergono contraddizioni sulla politica estera, una politica estera ondivaga, diversa da quella del precedente Governo, laddove si devono assumere grandi responsabilità istituzionali, quali l'approvazione del decreto‑legge di proroga della nostra missione di pace in Afghanistan, sul quale il Governo mesi or sono, per ottenere l'approvazione dal Parlamento, è stato costretto ad imporre la fiducia ai propri parlamentari dissidenti. il «no» dei tre Ministri recentemente dato nel volgere della seduta del Consiglio dei Ministri sul rifinanziamento della missione di pace in Afghanistan - tre Ministri del Governo si sono alzati e non hanno votato un decreto del proprio Governo - e le marce dei Ministri, che sicuramente verranno attuate da qui al 17 febbraio in occasione della protesta contro l'ampliamento della base di Vicenza. Il 17 febbraio vedremo Ministri del Governo Prodi, dinanzi alla dichiarazione del proprio Ministro della difesa che dà l'assenso all'ampliamento della base, marciare a Vicenza contro il loro Governo. quindi allo scenario di oggi che è estremamente grave e significativo.

impegno estremamente semplice e politicamente significativo, quello di «confermare che la politica estera italiana resta saldamente ancorata all'Unione europea, all'Alleanza atlantica e alle Nazioni Unite» istituzionalmente preposte che la scelta del Governo italiano di non opporsi all'ampliamento della base di Vicenza è, in primo luogo di rango politico e rientra nel quadro dell'appartenenza dell'Italia all'Alleanza Atlantica, nel rispetto degli accordi internazionali che ne derivano». è quel che chiedevamo e chiediamo nella nostra mozione e su questo chiediamo che l'Aula si pronunzi. Qual è la nostra politica? È una politica di continuità, come dichiara il ministro Parisi? Allora nelle dichiarazioni del ministro Parisi troviamo la condivisione di questo impegno chiesto al Governo. invece una politica diversa, di allontanamento dall'Alleanza euroatlantica, lo si dica in quest'Aula. Eravamo chiamati a votare questa mozione

accampare giustificazioni per noi insoddisfacenti. Questa è una mozione che è in piena sintonia con le parole del ministro Parisi e da qui discende la condivisione dell'ordine del giorno del centro‑destra, che condivide e approva la relazione del Ministro. Signor Presidente, posso non condividere la posizione della maggioranza - e della collega Finocchiaro - quando si sostiene che dietro questo ordine del giorno vi sia un atteggiamento strumentale dell'opposizione;

la commedia degli equivoci continua, con un ordine del giorno della maggioranza, la quale conia l'espressione «prendere atto delle dichiarazioni di un proprio Ministro». Ma la contraddizione di queste ore tocca il massimo là dove il rappresentante del Governo, chiamato ad esprimere il parere sull'ordine del giorno che approva la relazione di un proprio collega,

Signor Presidente, signori del Senato e del Governo, come abbiamo inteso dal dibattito, la decisione sull'ampliamento della base militare di Vicenza chiama in causa due competenze di livello differente: quella del Governo sulle scelte di politica estera e militare e quella che è in parte del Governo, anzitutto come proprietario del demanio militare, e in parte maggiore del Comune o dei Comuni interessati in materia di urbanistica, infrastrutture, assetto del territorio e ricadute sull'occupazione e sul sistema sociale. Stamane, il ministro Parisi si è pronunciato, in sostanza, sulla prima decisione (quella tutta di competenza governativa) affermando di non essere contrario - il che, per effetto della doppia negazione, significa essere favorevole - a confermare la presenza in Italia della base americana, tenendo anche conto del fatto serio che, in caso di diniego dell'ampliamento, l'intera brigata sarebbe, con ogni probabilità, trasferita altrove. riteniamo ‑ che la decisione responsabilmente assunta dal Governo sia da condividere, nel quadro dell'alleanza che dal 1949 lega l'Europa al Nord‑America

La portata politica della decisione non sfugge a nessuno, ma credo che il modo più razionale per guardarla bene sarebbe quello di svestirla dagli opposti ideologismi del filoamericanismo e dell'antiamericanismo assunti come ideologie, nel senso attribuito al termine da un compianto e grande membro di questa Assemblea, il senatore Norberto Bobbio, che descriveva l'ideologia come sistema di valori utilizzati per influire sui comportamenti di massa. Certo, nei tragici fatti di questi anni, prima con l'attacco terroristico alle Twin Towers e poi con la spedizione americana in Iraq, gli opposti ideologismi hanno avuto anche troppe ragioni per farsi valere. Rievocarli, però, non servirebbe a trovare la soluzione per la base di Vicenza, ed è apprezzabile che il dibattito, almeno fino alle penultime fasi, non vi abbia fatto troppo ricorso. La scelta che va oggi confermata è la decisione del Governo di autorizzare l'ampliamento della base americana sull'area del demanio militare, forse e possibilmente solo sul demanio militare, per non precludere ulteriori scelte urbanistiche da parte del Comune sulle aree restanti. Le installazioni americane in Italia sono un dato che risale alle origini della Repubblica, un elemento determinante dell'assetto difensivo del Mediterraneo e, non è il caso di tacerlo, un elemento decisivo nei rapporti attuali tra il Governo italiano e quello americano. A proposito di antiamericanismo ideologico, converrebbe guardarsi anche e soprattutto dalla sua rappresentazione antropomorfica che identifica l'America con la fotografia del suo Presidente *pro tempore*:

una collaborazione per la sicurezza, dove è minacciata, e per la costruzione della pace, dove non c'è. La politica estera italiana ha tre punti cardinali di orientamento: la politica comune europea, anche nel campo della difesa, la nuova missione dell'Alleanza Atlantica, rivolta principalmente al contenimento del conflitto e delle tensioni in Medio Oriente e, infine, il nuovo multilateralismo affidato all'organizzazione delle Nazioni Unite. Signori senatori, nessuno di quei tre riferimenti è realisticamente perseguibile se non si instaura un rapporto di nuova fiducia, di ritrovata parità politica, di multilateralismo efficace tra l'Europa, l'Italia e gli Stati Uniti. Certamente l'unificazione della Brigata americana sulla base di Vicenza, comporta - e l'interpellanza a firma della senatrice Pisa e di altri colleghi tocca giustamente il punto - il consenso da parte italiana per operazioni militari che partano dalla 173a Brigata. Non ho dubbi che il Governo italiano non si discosterebbe, nel caso, dalla corretta interpretazione degli accordi già fatti valere nelle circostanze precedenti (e se fosse qui il presidente Ciampi potrebbe dirci qualcosa in proposito), interpretazione da richiamare per la natura indiscutibilmente difensiva del Trattato Atlantico e dei *memorandum* conseguenti. Questo credo sia il merito del voto odierno del Senato che lascia aperte le fasi successive in cui si dovrà tener conto delle comprensibili preoccupazioni e delle legittime aspettative della cittadinanza vicentina. È di certo possibile ed opportuno che il Governo faccia la sua parte per concordare con gli enti locali le giuste contropartite, a cominciare dall'esonero delle amministrazioni locali dai costi infrastrutturali, dalle possibili cessioni di aree per servizi e spazi pubblici alle prospettive di occupazione. C'è un'opinione pubblica con cui, sempre nell'ottica dei buoni rapporti tra Italia e Stati Uniti, è obbligatorio fare i conti: il consenso che diamo alla decisione del Governo è anche un impegno in questo senso, formalizzato nell'ordine del giorno dei Capigruppo della maggioranza, con prima firmataria la senatrice Anna Finocchiaro. È escluso, per il principio di non contraddizione, il voto in favore delle mozioni presentate dall'opposizione, che pur contengono considerazioni e motivazioni anche apprezzabili, dietro le quali, peraltro, traspare, nei confronti del Governo, un atteggiamento di sfiducia e sospetto che, senatore Mantica, diventa esplicito proprio nella mozione presentata dove si arriva a parlare di Governo pregiudizievole per il prestigio internazionale del nostro Paese. Francamente non mi pare che le misurate comunicazioni del ministro Parisi meritino sfiducia e sospetto. Certo, tra le coalizioni, e anche all'interno di esse, le differenze ci sono, e come, non si tratta di occultarle, ma di metterle a confronto. Esercizio che, se non altro, avrebbe il vantaggio di indurre ciascuno a moderare l'orgoglio delle proprie certezze per arrivare, infine, ad un risultato che produca in positivo un effetto concreto. Il risultato consiste nell'ordine del giorno già richiamato, che prende atto delle comunicazioni del Governo - questo è un punto chiaro nella vicenda - e che nell'interesse delle popolazioni locali promuove la Conferenza già in programma per le servitù militari. Mi sembra un atto di consenso non enfatico, ma più attendibile rispetto all'inatteso entusiasmo dell'opposizione che approva con un ordine del giorno di sette parole le comunicazioni del Governo dopo aver dedicato quattro ore a criticarlo. Mi perdonerà il senatore Buttiglione se dico che mi ha fatto tornare in mente i banchi della scuola media, dove ci insegnavano "*timeo Danaos et dona ferentes*". Non è il caso di aprire le porte di Vicenza al cavallo di Troia. Abbiamo fiducia che, per la sincerità e lealtà del consenso che riceverà, il Governo uscirà rinfrancato da questo difficile scrutinio.

Signor Presidente, io non ho fatto delle scuole "pese", come diciamo noi, ma perlomeno siamo fuori tema con il nostro ordine del giorno. Dobbiamo discutere la questione della base di Vicenza e invece parliamo di altro. Prodi ha messo un treno, sul quale siamo saliti tutti, su un binario sbagliato sbagliato e l'ordine del giorno stabiliamo che tra un po' di tempo si farà una Conferenza sulla sicurezza dei trasporti. Ma che ci «azzecca»? O diciamo sì a Vicenza o diciamo no a Vicenza. caso, credo che chi dice di essere comunista, chi socialista, chi democratico (italiano, perché i democratici americani pare che vogliano ridiscutere la politica di guerra americana) dovrà pur cominciare a interrogarsi,

nel Paese non cresce la fiducia nella classe dirigente e nelle forze politiche. Dire una cosa fino a Vicenza e poi farne delle altre non è chiaro, non è una politica.

dell'Unione su quel programma, sulle scelte sbagliate no. La responsabilità non è nostra se oggi arriviamo a questa discussione. Quindi, se anche si fosse fatto il "copia e incolla" con l'articolo 11 non c'entra niente con la discussione di Vicenza.

che ad essa è affidata la sorte del Governo. Quali parole sono state dette oggi in questa sede? Vorrei ricordare due cose. Quando si esprime al Governo si scrivono ordini del giorno di questa natura. Cito l'ultimo del 19 maggio, quando è stata espressa la fiducia al Governo Prodi "Il Senato della Repubblica, udita la relazione del Presidente del Consiglio dei ministri, esprime la fiducia al Governo e passa all'ordine del giorno".

il Governo è contrario a questo nostro ordine del giorno. Cosa accade dal punto di vista istituzionale se il Senato boccia questo ordine del giorno? C'è ancora la fiducia al Ministro? C'è la fiducia a questo Sottosegretario che in Aula invita a votare contro il Governo o ci sono altre conseguenze? Quanto vale la presa di posizione del Senato in questo momento, come Parlamento, nei confronti del Governo?

In questa sede facciamo le leggi, scriviamo questioni cogenti. Quello che viene detto qui vale per tutto il Paese. Chi trasgredisce queste regole alcune volte va in galera (prima che ci fosse l'indulto, ora non più).

in questo caso, dell'opposizione. Se invece l'ordine del giorno viene approvato e c'è la fiducia verso il Governo, la fiducia verso il Governo, credo che l'ordine del giorno presentato dai Gruppi della maggioranza, oggi diventata opposizione, non dovrebbe comunque essere votato perché

Abbiamo un articolo del Regolamento che esplicitamente affronta il problema e lo risolve. Ci saranno state delle ragioni per decidere esplicitamente. Molte cose si fanno con riferimento ai precedenti. La votazione sulle mozioni ha la precedenza su quella degli ordini del giorno che le concernono. Questo dato esplicito del Regolamento non consente aggiustamenti. La questione posta dal senatore Castelli è invece molto delicata. Gli atti del Senato sono atti ufficiali e non c'è dubbio che siano tutti carichi di conseguenze politiche.

abbiamo assistito questa mattina alle dichiarazioni del ministro Parisi, che credo non possa non condividere le proprie dichiarazioni. Il Vice ministro esprime parere contrario su un ordine del giorno in cui si approvano

richiamo regolamentare è all'articolo 72 del Regolamento: se un Vice ministro esprime parere contrario alle dichiarazioni di un Ministro, o sta oltraggiando il Governo, e si dimette, o sta oltraggiando il Senato, e lo ha fatto questa mattina. Le chiedo, signor Presidente, perché l'articolo 72 lo prevede, e mi spiace che se ne sia andato, ma chi oltraggia il Senato deve essere arrestato in Aula.

un giudizio politico su tutto l'andamento dei lavori, ma che qualcosa che lei giudica una contraddizione possa essere un oltraggio questo non risulta né dall'articolo 72, né da altri punti del Regolamento.

Presidente, l'ordine del giorno G3 è precluso. Non può essere messo in votazione, è assorbito dal voto che che approva la relazione! È precluso, signor Presidente! Non può lei mettere in votazione questo ordine del giorno perché è precluso! È precluso dalla logica!

né mi consentirò espressioni che pur ho sentito risuonare in quest'Aula. Voglio dire una cosa molto semplice. Ho detto che non lo faccio, mi dispiace che il mormorio arrivi da chi l'ha fatto. Non c'è dubbio che ci troviamo di fronte alla vittoria politica del centro-destra sull'ordine del giorno che strumentalmente dà fiducia al Governo per il tramite di una presa d'atto favorevole delle comunicazioni del Ministro. questa situazione è tanto imbarazzante per il centro-sinistra quanto lo è per il centro-destra. Tuttavia, siccome voglio andare alla natura e alla sostanza politica della questione e della nostra difficoltà - se mi fate parlare - dovrei dovrei dire che chi fosse un osservatore attento, e non mi fermo soltanto ai simboli, dovrebbe prendere atto che in questi giorni sui giornali e stamattina con dovizia di argomenti, tutti legittimi naturalmente, adoperati dai colleghi del centro-destra, l'operato del Governo Prodi in materia di politica estera è quanto di più dannoso, devastante - come ha detto la collega e pregiudizievole, rispetto alle relazioni tra il nostro Paese e la comunità internazionale, che si possa immaginare. Più volte è venuta dai banchi del centro-destra la necessità di mettere un freno alla devastante azione del Governo Prodi e, dunque, più volte si è alzata dai vostri banchi la protesta. Ora è ovvio che l'ordine del giorno che avete presentato è del tutto strumentale, così come è ovvio che le argomentazioni adoperate dal presidente Matteoli Matteoli sono fortemente impressive dal punto di vista politico, ma che non possono avere nessun pregio sotto il riguardo della questione istituzionale poiché la questione di fiducia è regolata dalla Costituzione e dalla legge e poiché, come è fin troppo ovvio, questo voto, per quanto riguarda la tenuta del Governo, non ha alcuna possibilità di incidere sulla valutazione della tenuta della maggioranza. il fatto di rifiutare la possibilità di avere un voto sulla mozione che vede le firme di tutti i Capigruppo di maggioranza diventa a questo punto un ulteriore ostacolo frapposto a questa verifica. verifica. So che in Aula i numeri che poco fa abbiamo registrato pongono una questione politica. Quindi, vorrei essere molto chiara con i colleghi: non la sto archiviando e non sto mettendo la polvere sotto al tappeto perché è ovvio che questo voto rappresenta per noi, per i tanti o per i pochi, che anche nel mio Gruppo non hanno votato Brava!),* la necessità di una assunzione di responsabilità. Vi dico anche che allo stesso modo vorrei che i componenti della coalizione dell'Unione riflettessero riflettessero sul fatto che se ci fossimo astenuti dal votare questo risultato non si sarebbe prodotto. Ma quel che voglio dire è che se intatta è la questione politica che viene fuori dal voto di oggi, ciò che mi pare assolutamente improbabile e sotto il profilo istituzionale e politico del tutto improponibile è che questa vittoria del centro-destra di oggi abbia un riflesso, uno soltanto, sulla vicenda che riguarda la tenuta del Governo Prodi e la sua possibilità di legittimamente governare. Questo è francamente argomento che capisco viene giustamente adoperato; lo avremmo fatto pure noi, colleghi, con la stessa e forse con più aggressiva forza questo è argomento che purtroppo ha la caducità di questo passaggio di minima cronaca.

con una dichiarazione del Presidente e con l'approvazione della relazione del Ministro della giustizia, abbiamo votato tutti gli i documenti "Conformemente..." - ha dichiarato il Presidente prima del voto - "alla prassi del Senato, le proposte di risoluzione saranno poste ai voti secondo l'ordine di presentazione, con l'intesa che l'esito di ciascuno dei voti non sarà ostativo alla votazione delle risoluzioni successive che si intenderanno messe ai voti per le parti, eventualmente, non precluse, né assorbite". Questa è la prassi che il 24 gennaio abbiamo seguito. Inoltre, i due ordini del giorno formalmente non si contraddicono e vi è una prassi rigida del Senato. Di cosa stiamo discutendo? La cosa politica è un fatto; il fatto procedurale è un altro. Quindi, metterò ai voti l'ordine del giorno, sulla base di queste regole. Possiamo anche discutere duramente su tutto il resto, ma perché sciupare l'ordine di un dibattito di grande valore politico,

sull'intervento della senatrice Finocchiaro, ma, per economia dei lavori, le dichiaro soltanto la mia solidarietà per aver dovuto affrontare un momento così difficile. Sa anche lei che ha dovuto arrampicarsi sui vetri! Ma, Presidente, vi è una questione fondamentale. Lei ha citato un precedente; ebbene, vi sono centinaia e centinaia di precedenti che dichiarano preclusi i documenti che vanno in senso contrario rispetto a quello approvato. Vorrei ricordare che qui c'è stato un parere preciso del Governo, che ha espresso un parere favorevole sul documento della sinistra e un parere contrario su un documento della Casa delle Libertà. Quindi, non è vero che i due documenti non sono l'uno contro l'altro. Pertanto, è del tutto evidente che in questo caso, per una prassi consolidata del Senato, questo voto assorbe quello successivo, perché c'è stato un parere preciso del Governo. Se il Governo si fosse rimesso all'Aula, capirei allora la sua posizione. Per quanto ci riguarda, il Gruppo della Lega Nord non parteciperà a nessuna altra votazione, perché il Senato si è espresso chiaramente.

ho ascoltato con attenzione e ho preso atto delle dichiarazioni della collega Finocchiaro. È innegabile che lo stato di disagio del centro-sinistra non può essere paragonato a quello del centro-destra, per il semplice fatto che nel centro-destra non c'è nessun disagio, anzi, vi è la consapevolezza che questo voto dell'Aula ha consegnato alla storia un dato: in questo momento, il Governo Prodi non ha una maggioranza parlamentare sulla politica estera. Si pone un problema di legittimità a continuare a governare o meno, è un problema politico, un problema sul quale auspichiamo l'autorevole attenzione e l'eventuale intervento del Presidente della Repubblica. È un Governo che già era in crisi un'ora fa, quando attraverso un suo esponente aveva dato un parere contrario ad un ordine del giorno che approvava la relazione di un Ministro. Già la crisi era nei fatti, lo avevamo detto nel nostro precedente intervento; adesso si è consolidata con il voto liberamente espresso da questa Aula.

perché non vi è una presa d'atto, vi è una condivisione dell'Aula della relazione del rappresentante del Governo, non certo una presa d'atto. *(Applausi dal Gruppo FI)*. Quindi, quella dichiarazione Allora, per rispetto al precedente voto, annunziamo che, ove ella, nella sua autonomia, dovesse ritenere di mettere ai voti l'ordine del giorno che reca la prima firma della collega Finocchiaro, non parteciperemo al voto, per il semplice motivo che riconosciamo che ormai si è consumato in quest'Aula un dato politico, la crisi di un Governo, ed è perfettamente inutile votare su un documento che è stato già implicitamente bocciato dal precedente voto. Quindi, come Forza Italia e ritengo come centro‑destra, non parteciperemo al voto; questo ordine del giorno se lo approvi una maggioranza che non è più tale in quest'Aula del Senato. voglio fare una pacata riflessione. Rispetto alle sue considerazioni e alla sua tesi, il rispettare precedenti vicinissimi e mettere ai voti un altro ordine del giorno, ove fosse approvato, non stravolgerebbe il voto che già c'è stato. Io faccio rispettare una regola.

Vi prego di stare a questa considerazione.

tale, e si voti per parti separate. Noi non abbiamo niente in contrario alla conferenza sulle servitù militari. Noi voteremo contro la prima parte, se messa in votazione, e a favore della seconda, se la votazione avviene per parti separate. Se invece si insiste sulla votazione unica, ce ne andiamo tutti perché evidentemente è clamoroso l'errore della maggioranza.

Qui non siamo davanti ad un semplice ordine del giorno (che, tra l'altro, se accolto dal Governo potrebbe non essere neppure messo in votazione), ma ad un fatto politico su cui il Governo deve riflettere, perché il Governo oggi ha una maggioranza, ma non è quella che gli ha dato la fiducia sulla politica estera.

che non è possibile passare alla votazione dell'ordine del giorno di cui è prima firmataria la collega Finocchiaro.

che lei possa cercare, con gli Uffici, una scappatoia politica in un momento così delicato, ma, almeno su questo, credo che lei non possa darci torto. La prima parte è preclusa; a nostro avviso,

con la prima parte, che è però sicuramente preclusa. Non c'è costituzionalista o giurista che possa sostenere il contrario, nemmeno arrampicandosi sugli specchi come lei sta cercando di fare in questo momento come Presidente. C'è anche un altro aspetto

Comunque sia, la prima parte non può essere messa in votazione. Se lei insiste, signor Presidente, noi siamo costretti ad abbandonare l'Aula perché non possiamo subire questo. È assolutamente inaccettabile. *(Applausi dai Gruppi

Matteoli, la prima regola di ogni Assemblea democratica è che le votazioni si svolgano nell'ambito di un procedimento nettamente limpido e chiaro. La prima regola è che, individuato un percorso, questo percorso venga rispettato. Presidente, all'inizio dei nostri lavori, la Presidenza dell'Assemblea, senza alcuna contestazione, ha annunziato che le mozioni e gli ordini del giorno sarebbero stati tutti votati e che nessuna approvazione avrebbe precluso le votazioni successive. Presidente, è del tutto evidente ‑ e mi spiace che i colleghi dell'opposizione tergiversino ‑ che il comportamento della maggioranza si è uniformato a questa comunicazione del Presidente dell'Assemblea; noi, cioè, abbiamo votato sapendo che non vi sarebbero state preclusioni. Ora le preclusioni non possono intervenire in corso d'opera. signor Presidente, fatta questa affermazione di principio e di legittimità dei nostri comportamenti, se può essere di aiuto

anche perché prendere atto della relazione del Governo e del Ministro, in qualche modo, per una certa parte, significa anche condividerla. Quindi, non abbiamo difficoltà, atteso che in quest'Aula una maggioranza,

così dire ‑ per favorire la prosecuzione dei lavori, ma il principio è che abbiamo votato nell'ambito di un procedimento certo e non possiamo essere essere danneggiati nei nostri comportamenti per una modifica di questo procedimento. Accettiamo la soluzione per trovare un modo comune di andare avanti, ma le nostre ragioni sono indiscusse.

dal precedente del 24 gennaio scorso, perché è questo il modo di operare del Senato. Se il senatore Boccia dice che la che la maggioranza è disposta a ritirare la prima parte del provvedimento e quindi ad eliminare il giudizio sulle comunicazioni del Governo, questo scioglie anche la difficoltà che voi state sottolineando, perché restano un ordine del giorno che approva

Dopodiché, si vuole una conferenza? Ciò è un po' irrituale, perché non se n'è mai parlato nel dibattito (si è parlato di tutt'altro), tuttavia, perché negare una conferenza? *(Applausi del senatore Storace)*. Noi siamo interessati ad una conferenza che approfondisca questi problemi e voteremo a favore.

esegetico. È ovvio che la premessa: «Preso atto delle comunicazioni del Governo e del dibattito aperto tra le forze politiche e l'opinione pubblica» è un *incipit* che ha un senso politico. Tale senso politico si trova riprodotto, identicamente, nella seconda parte dell'ordine del giorno, che come sapete è copiata dal programma dell'Unione, dove si dice «al fine di arrivare ad una soluzione condivisa che salvaguardi al contempo gli interessi della difesa nazionale e quelli, altrettanto legittimi, delle popolazioni locali».

positiva sviluppi un impegno a salvaguardia e in considerazione degli altrettanto legittimi interessi delle popolazioni locali.

strettamente esegetico parlamentare, perché rischieremmo di amputare un'affermazione politica, la nostra ovviamente, che ha un valore

È emerso precisamente che sono minoranza su questioni rilevantissime di politica estera e stanno cercando, in tutti i modi, di uscire da quest'Aula con un voto favorevole sul loro documento. Ora, siccome è importantissimo

è inammissibile: parla di tutt'altro e non c'entra nulla con l'ordine del giorno. Io e il mio Gruppo a questo giochetto non ci stiamo e abbandoniamo l'Aula.

però, anche una di carattere logico: non si può prendere atto di un qualcosa che si è già approvato, perché se n'è già preso atto per poterlo approvare; la presa d'atto successiva all'approvazione dimostrerebbe, quindi, un dato di schizofrenia istituzionale del Senato e non di coerenza politica.

Non vi era nulla di strumentale in ciò, perché la nostra posizione è a favore dell'ampliamento della base di Vicenza: questa posizione ha espresso il Governo e questa noi abbiamo votato.

contrario: è un fatto politico ineludibile ed il silenzio glaciale di un Governo sfiduciato dalla propria maggioranza ne è testimonianza.

I precedenti della storia parlamentare hanno visto Governi rassegnare le dimissioni in poche ore; inoltre, non possiamo votare altro perché il Senato si è espresso per ragioni politiche, senza alcuna strumentalità.

gennaio: «Conformemente alla prassi del Senato, le proposte di risoluzione saranno poste ai voti secondo l'ordine di presentazione con l'intesa che l'esito di ciascuno dei voti non sarà ostativo alla votazione delle risoluzioni successive che si intenderanno messe ai voti per le parti, eventualmente, non precluse, né assorbite». Vi è un discorso di questo genere: altre volte abbiamo votato, qual è il grande ostacolo che ci impedisce di farlo ora?

Se qualcuno, anziché votare a favore di un ordine del giorno che approvava le dichiarazioni del Governo, ha preso una cantonata volendo che si votasse contrario, non può adesso far rientrare dalla finestra

così. Qui non si può sovvertire un'interpretazione, perché le parole scritte in questo precedente sono assolutamente chiare. Ciò non toglie nulla alla forza di una decisione politica assunta dal Parlamento.

ad impiccarci con le frasi e le virgole, perché se pensate, come sosteneva il collega Castelli, che con un voto successivo si possa ribaltare

abbia un significato politico talmente elevato da consentire a me di chiederle, Presidente, di sospendere la seduta, in attesa che il Governo ci faccia conoscere la linea di politica estera che intende adottare per il Paese, visto che è stato

ho pieno rispetto delle conclusioni politiche, e sottolineo politiche, che i colleghi dell'opposizione hanno dato

al dibattito aperto tra le forze politiche e nell'opinione pubblica, volendo, e votando, che il Governo si impegni ad organizzare una conferenza sulle servitù militari. È questo che vuole il Paese, signor Presidente, colleghi. Non nascondiamoci dietro un dito. Voi avete votato e noi abbiamo votato contro l'ordine del giorno Calderoli in quanto strumentale. Avete raggiunto il vostro fine; va bene, lo si accetta. La destra ha appoggiato la linea politica del Governo; la appoggiamo anche noi, però, andiamo oltre. Vogliamo che si avvii questa conferenza e chiedo a questo ramo del Parlamento

Signor Presidente, io credo che sia nell'interesse di tutti evitare che il significato politico di un voto venga travolto da una contesa dubbia su questioni procedurali. Non era un voto strumentale, senatrice Finocchiaro, e comunque nessuno qui ha titolo per dichiarare strumentale questo o altro l'ordine del giorno. Abbiamo semplicemente approvato le dichiarazioni rese dal Ministro, intendendo così approvare la scelta di autorizzare l'ampliamento della base di Vicenza. A questo voto legittimamente si è contrapposta la maggioranza di Governo. Ora, io credo che non sia ammissibile alcun voto che tenda a

frequento le Aule parlamentari - ahimè - dal lontano 1972 e non mi è mai accaduto di assistere ad un incidente di questo genere dopo il quale il Governo non abbia chiesto una pausa di riflessione per poter considerare l'accaduto e proporre all'Aula e alla sua maggioranza una valutazione appropriata.

si andavano a ricercare i precedenti di quando il Parlamento era ancora a Firenze. In una discussione, per aggirare una proposizione che non si voleva far discutere, si citò un'abile mossa di un deputato al Parlamento di Firenze, quando si cercava di confondere la Questione Romana con problemi di carattere politico, che fece approvare un bellissimo ordine del giorno: "Il Parlamento, nulla curandosi dell'infallibilità pontificia, passa all'ordine del giorno". Oggi noi abbiamo avuto una novità. La novità che da anni abbiamo introdotto un'interpretazione nella Costituzione sul voto di fiducia

Adesso siamo dinanzi ad una innovazione, perché il voto di fiducia è venuto su una proposizione dell'opposizione. Comunque, è venuto: cioè, si è creata la possibilità

Io, anche nella consapevolezza che, rispetto alle tesi sostenute da esponenti del centro-destra, la dizione del precedente a cui mi riferisco non mette in discussione le considerazioni politiche svolte,

Ho corretto la votazione con la mia scheda, ma, nonostante abbia estratto la scheda del senatore Baccini, il voto è stato registrato ugualmente, nonostante la mia segnalazione alla Presidenza. Probabilmente, la Presidenza aveva già chiuso la votazione.